Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche al calendario della settimana corrente nonché il nuovo calendario dei lavori fino al 24 marzo. Fermi restando gli argomenti già previsti, il calendario della settimana corrente è integrato con la discussione del decreto-legge sulla festa nazionale del 17 marzo 2011, ove concluso dalla Commissione. Il calendario della prossima settimana prevede, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, la discussione del disegno di legge recante modifiche al codice di procedura penale a tutela del rapporto

I Presidenti dei Gruppi di opposizione sono stati invitati a indicare i disegni di legge fatti propri dai Gruppi medesimi, ai fini di un prossimo inserimento nel calendario dei lavori. Infine, con riferimento all'esame presso la Commissione affari costituzionali dei disegni di legge in materia elettorale, il Presidente ha richiamato l'attenzione dei Capigruppo circa l'esigenza, manifestata dal Presidente della Commissione medesima, che sulla materia siano presentate iniziative proprie dei Gruppi.

Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il disegno di legge che oggi presentiamo al voto dell'Aula riguarda la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate nei mercati regolamentati e trae origine dal testo già approvato alla Camera dei deputati al quale, qui in Senato, si erano affiancate altre iniziative di legge. Sulla materia si è detto e si è scritto molto, ma soprattutto voglio ricordare oggi in Aula che a questo tema sono stati dedicati gli interventi delle tre più alte cariche dello Stato il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato e il Presidente della Camera - che hanno toccato, in occasione dell'8 marzo, lo specifico argomento delle quote rosa negli organi di governo e, più in generale, la parità tra donne e uomini nella nostra società. Tra tutti, voglio ricordare le parole del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per il quale «il grado di impegno delle donne per affermare la parità è tra i principali indicatori della maturità e dello stato di salute dei sistemi democratici». Secondo il Presidente della Repubblica, «le donne italiane sono lontane dal raggiungimento della parità in vari campi». Dal 1861, ha ricordato il Capo dello Stato facendo un *excursus* storico, «è stato fatto un lungo cammino, le donne hanno progressivamente conquistato spazi e diritti, con una forte accelerazione nell'ultimo cinquantennio». Tuttavia, il divario di genere risulta anche dai rapporti internazionali, nella rappresentanza politica, nei *media*, ancora in qualche carriera pubblica, nella conduzione delle imprese e si manifesta anche nell'accesso al mercato del lavoro. «Per raggiungere una parità sostanziale tra uomo e donna», secondo il Capo dello Stato, «è necessario incidere essenzialmente sulla cultura diffusa, sulla concezione del ruolo della donna, sugli squilibri persistenti e capillari nelle relazioni tra i generi, su un'immagine consumistica che la riduce da soggetto ad oggetto, propiziando comportamenti aggressivi(...)». Parole esplicite e molto eloquenti. Perché, se è vero che in Italia è costituzionalmente prevista l'affermazione del principio di pari opportunità, è ancora più vero che essa è continuamente aggirata, come dimostrano tutti gli indicatori: rappresentanza di genere nelle istituzioni pubbliche, dirigenza nelle imprese, nella vita politica e nei partiti, livelli di occupazione. A livello mondiale il *trend* ha subito, già da diversi anni un'inversione di tendenza: le donne sono talmente al centro della vita politica ed economica, tanto che è stato coniato il termine *womenomics*, che descrive il ruolo sempre più importante che esse stanno interpretando e continuano ad interpretare nella vita economica.Quindi, donne che prendono decisioni, donne che hanno anche più cultura e maggiori potenzialità di guadagno delle loro madri, donne che con i loro investimenti hanno un impatto economico determinante e si avviano a costituire la forza trainante dell'economia globale. È questo il nuovo mondo femminile al quale deve porre attenzione la politica, al quale deve guardare chi si preoccupa di garantire pari opportunità. donne al vertice delle imprese italiane sono poche, molto meno della media europea e questo è un fenomeno noto, di cui da qualche tempo si é iniziato a discutere. Secondo le statistiche della Commissione europea, l'Italia è al ventinovesimo posto, su trentatré Paesi censiti, per numero di donne presenti nei consigli d'amministrazione delle società quotate in Borsa, seguita solo da Malta, Cipro, Lussemburgo e Portogallo.

la Norvegia ha inserito l'obbligo, dal 1° gennaio 2006, per le società quotate alla Borsa di Oslo di riservare alle donne una parte

è arrivata dopo un periodo di prova di due anni, nel corso dei quali le società avevano la possibilità di ottemperare volontariamente. Ma prima di affrontare il nostro argomento all'ordine del giorno, cioè la rappresentanza femminile negli organi di governo, desidero qui ricordare ciò che lo stesso Presidente del Senato, Renato Schifani, ebbe a dire il 14 febbraio scorso, annunciando che avrebbe senza indugi calendarizzato in Aula il nostro disegno di legge. L'annuncio, molto significativo, avvenne in contemporanea alla presentazione del neo Segretario generale del Senato, dottoressa Elisabetta Serafin, la prima donna a ricoprire tale prestigioso incarico. Le pari opportunità sono un'espressione ormai molto diffusa ed un concetto giuridico-politico che si è affermato in molti settori della nostra società ed anche nella sensibilità individuale di ciascun cittadino, In altri termini, le pari opportunità non sembrano trovare più gli oppositori di un tempo e vengono, almeno in teoria, sottoscritte da tutti. C'è però, come spesso avviene, un'abissale differenza tra le parole e i fatti. Ed è allora necessario intervenire, caso per caso, e rendere operativo quel principio giuridico-politico di cui si parlava. Ed è con tale criterio che è nato il disegno di legge al nostro esame. La classifica relativa alla presenza femminile sul *Gender Gap* del World Economic Forum ha evidenziato un peggioramento dell'Italia. Nel nostro Paese, infatti, sono particolarmente penalizzati l'accesso e le opportunità delle donne proprio nel mondo del lavoro. Eppure le statistiche dimostrano che le donne riescono meglio negli studi, si laureano prima e con voti superiori rispetto agli uomini. considerando lo stipendio come uno dei parametri di valutazione delle pari opportunità in tutti i campi, le donne *manager* in particolare, guadagnano circa il 12 per cento in

*relatrice*. E un dato ancora più sconfortante è legato alla maternità: tre donne *manager* su quattro non hanno figli. Per le donne lavoratrici, la situazione non è certo migliore, anzi in certi settori produttivi peggiora vistosamente. È forse il caso di chiedersi quanto ciò dipenda da una scelta volontaria, oppure se si tratti di una scelta indotta da un contesto sociale poco orientato alla valorizzazione delle donne. Per questo è necessario mettere in campo ogni utile iniziativa, compresa l'introduzione di una norma di garanzia che assicuri l'equilibrio tra i generi. Perché includere sempre più donne nel mercato del lavoro non vuol dire favorire soltanto le donne, ma favorire nel suo complesso tutto il Paese, che non può permettersi di avere il 50 per cento di talenti femminili inutilizzati. Non a caso, in America, l'8 marzo è definito Giornata internazionale di azione delle donne. Una differenza non solo terminologica che testimonia un diverso approccio culturale, sicuramente più pragmatico e meno retorico rispetto a quello italiano. Quest'anno l'8 marzo per tutti gli italiani ha assunto però una connotazione davvero unica e diversa rispetto al passato, alla luce delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, per la quale tante donne si sono battute. credo che sarebbe importante prevedere iniziative specifiche sul ruolo che le donne hanno svolto per l'Unità d'Italia: la loro eroica partecipazione al Risorgimento nazionale e la loro eroica partecipazione, anche nel corso de**l** XX secolo, a

Sulla rappresentatività femminile nel Parlamento dobbiamo conclusivamente ricordare una nota positiva. Con le elezioni del 2008 si è raggiunto il miglior risultato di rappresentanza femminile: 110 donne elette alla Camera dei deputati e 46 al Senato della Repubblica. Se il conseguimento della percentuale paritaria del 50 per cento per le donne elette in Italia sembra essere un traguardo ancora troppo ambizioso da raggiungere, vi è tuttavia un elemento che può essere interpretato come disaffezione

Se si osservano i dati, anche solo per quanto riguarda le ultime tornate dopo la riforma elettorale del 1993, può essere constatato un progressivo aumento dell'astensionismo in generale, e in particolare di quello femminile, che non viene più considerato come l'esito di un processo di socializzazione improntato sul modello maschile, quanto piuttosto la conseguenza di un fenomeno collegato all'effetto centro-periferia, secondo il quale le donne partecipano meno alle elezioni perché si trovano ad una maggiore distanza

Prima di passare alla disamina del testo, per la quale rimando alla relazione introduttiva all'articolato, va detto che durante la discussione in Commissione finanze sono emerse alcune criticità sul testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, che sono state attentamente analizzate e hanno permesso di giungere ad un testo condiviso. Pertanto, a partire dal 14 febbraio e fino al 10 marzo, si è svolto in Commissione, qui a Palazzo Madama, un lavoro legislativo molto intenso e molto proficuo che ha consentito di superare non pochi ostacoli e giungere alla condivisione di un testo che rappresenta un giusto equilibrio tra le istanze del mondo femminile, il testo che ci è giunto dalla Camera dei deputati e le sollecitazioni e richieste che ci sono state avanzate da chi rappresenta le società, da chi rappresenta le industrie, da chi rappresenta il sistema bancario e finanziario del nostro Paese. I punti critici del testo pervenuto dalla Camera riguardavano, in particolare, la gradualità delle quote, il regime sanzionatorio e la disciplina delle società pubbliche. Il Governo dal canto suo ha presentato tre emendamenti che pure raccoglievano le sollecitazioni pervenute, ma che - a giudizio della Commissione - si discostavano troppo dal testo che ci era arrivato dalla Camera, in Camera, in particolare per ciò che riguarda la gradualità e il regime sanzionatorio. Quindi, è stato svolto un importante lavoro di sintesi e di mediazione tra il testo del Governo e i subemendamenti presentati, che ha permesso alla Commissione di licenziare un articolato condiviso. Di questo intendo ringraziare il vice presidente della Commissione, senatore Ferrara, che ha svolto un lavoro importante e meticoloso anche dal punto di vista del richiamo al Regolamento.

nei consigli di amministrazione e comunque negli organi di governo delle società quotate e delle società pubbliche (distinguo perché abbiamo anche dovuto

per le società pubbliche, in quanto non sottoposte e non soggette alla vigilanza della CONSOB).

tratta cioè di un regime transitorio. Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, il testo del Governo prevedeva l'applicazione della sanzione amministrativa, a differenza del testo pervenuto dalla Camera che prevedeva la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione nel caso in cui al primo rinnovo non si fosse raggiunta la quota del terzo. Anche qui credo che abbiamo trovato, insieme a tutti i Gruppi, un buon punto di sintesi. Il testo sul quale abbiamo convenuto prevede, nel caso in cui la società non si adegui a quanto previsto dalla legge, una

Il regime ovviamente cambia nel caso del collegio sindacale (è evidente, infatti, la diversa importanza: il consiglio di amministrazione è il cuore della società, il collegio sindacale, pure importante, è comunque un organo di vigilanza e controllo), in ordine al quale la sanzione amministrativa è inferiore, e va dai 20.000 euro ai 200.000 euro. Abbiamo inoltre previsto

Per quanto riguarda le società pubbliche che - come già detto - non rientrano nella vigilanza della CONSOB, è prevista l'emanazione di un decreto attuativo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, per disciplinare in maniera uniforme

sia stata riconosciuta la centralità del ruolo del Parlamento in quanto rappresentanza reale dei cittadini, e per questo voglio ringraziare il sottosegretario Viale.

dei senatori del Popolo della Libertà, Maurizio Gasparri, ha espresso grande soddisfazione in merito e ha sottolineato il proficuo lavoro svolto dalla Commissione in un clima di collaborazione tra maggioranza e opposizione. Ricordo poi l'importante dalla Presidente del Gruppo del PD, senatrice Anna Finocchiaro, grazie anche alla sua esperienza in materia in quanto primo Ministro delle pari opportunità della Repubblica italiana. Infine, ringrazio tutti i membri della Commissione finanze che sono intervenuti tutti quei senatori che hanno espresso il loro dissenso, avendolo fatto in modo costruttivo e presentando subemendamenti di cui abbiamo tenuto conto nel nostro lavoro. Da ultimo ringrazio il senatore Barbolini

senatori, prima di iniziare i lavori che porteranno quest'Aula ad esprimere il voto finale, che mi auguro arrivi con lo stesso spirito che ha contraddistinto le attività svolte presso la Commissione finanze, voglio ringraziare tutti i membri di questo ramo del Parlamento che hanno consentito di presentare un testo basato su una intesa tra tutti i Gruppi che hanno operato in sede redigente. Il testo che si vota oggi è il frutto di un confronto intenso e costruttivo per il raggiungimento di un accordo che rispettasse i principi ispiratori del testo licenziato all'unanimità in prima lettura alla Camera, ma che al contempo tenesse conto delle richieste di chi auspicava una maggiore gradualità di applicazione delle norme. Il dibattito sviluppatosi nella Commissione finanze è stato acceso, talvolta appassionato, ma sempre corretto e rispettoso delle diverse posizioni delle parti. Ritengo che il testo del disegno di legge licenziato dalla Commissione sia equilibrato e ragionevole e presenti importanti e significative novità rispetto al testo originario licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Sottolineo al riguardo la necessaria ed opportuna gradualità che è stata prevista prima di pervenire al provvedimento, che tuttavia spero non debba mai essere assunto, della decadenza degli organi di controllo e dei consigli di amministrazione per la mancata osservanza delle disposizioni oggi in esame. Così come, con riguardo alla composizione dei consigli di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate e delle controllate pubbliche non quotate, ritengo necessario sottolineare quanto la posizione assunta dal Governo in sede redigente sia stata di grande coerenza e responsabilità. Mi riferisco, in particolare, al parere espresso sulla proposta della relatrice di modificare l'emendamento del Governo relativo alla composizione dei consigli di amministrazione e degli organi di controllo che dovranno ora essere composti da un quinto del genere meno rappresentato a partire dal 2012 e da un terzo a Sul punto, voglio sottolineare come il Governo fosse sostanzialmente in linea con tale previsione fin da subito, avendo tuttavia proposto, con l'emendamento presentato, una maggiore gradualità temporale nel pervenire al medesimo risultato attraverso un passaggio ulteriore che stabiliva, in un primo momento, l'obbligo di adeguare i citati organi con una presenza del genere meno rappresentato di almeno un decimo del totale, arrivando solo successivamente all'obbligo di un quinto. Per tale ragione, e non quindi per una contrarietà preconcetta, che mai c'è stata, rispetto alla volontà dell'intera Commissione di non prevedere questo primo passaggio, anticipando da subito l'obiettivo di un quinto, il Governo ha ritenuto opportuno porre in essere ulteriori valutazioni necessarie a verificare l'impatto che tale risultato avrebbe prodotto nell'ambito di realtà societarie che, non dimentichiamolo, costituiscono in molti casi l'asse trainante della nostra economia. Anche nei Paesi dell'Unione europea il tema è particolarmente sentito. La comunicazione della Commissione europea del 21 settembre 2010 sulla strategia per la parità tra uomini e donne vede una correlazione positiva tra le donne in posizioni dirigenziali ed i risultati economici nelle società quotate. In questo quadro, il dibattito si concentra su quali siano le migliori modalità per assicurare un'adeguata presenza femminile negli organi di amministrazione e controllo. In Europa gli Stati membri percorrono strade diverse. Tra i Paesi nordici, la Norvegia ha già previsto da anni le quote rosa, mentre in Islanda queste saranno operative dal 2013. Anche la Spagna e la Francia hanno recentemente optato per un intervento regolatorio: in Spagna, entro il 2015 le imprese con più di 250 dipendenti dovranno approvare dei piani di equilibrio di genere, e le società più grandi dovranno riservare alle donne almeno il 40 per cento dei posti disponibili nel consiglio di amministrazione; quest'anno è stata approvata una legge che riserva al genere meno rappresentato il 20 per cento degli amministratori dal 2014, e il 40 per cento degli amministratori dal 2017. In Germania, non volendo per ora prevedere l'introduzione per legge delle quote rosa, è stato reso più stringente il codice di regolamentazione societaria. Infine, nel Regno Unito si raccomanda di assicurare entro il 2015 una presenza femminile pari ad almeno il 25 per cento degli amministratori. Nel valutare la soluzione più idonea per l'Italia, non può essere trascurato che il nostro Paese presenta un esiguo numero in percentuale di donne ai vertici aziendali. Nella recente analisi sull'attuazione del codice di autodisciplina riferita all'anno 2010, appena resa pubblica da Assonime, si legge che le donne presenti nei consigli di amministrazione rappresentano il 6 per cento del totale, mentre le donne presenti nei collegi sindacali sono il 7 per cento Sembra quindi appropriata una azione legislativa temporanea - sottolineo, temporanea - capace di imprimere un'accelerazione alla presenza femminile negli organi di amministrazione e controllo, altrimenti difficilmente realizzabile, ferma restando la gradualità nell'applicazione della misura, al fine di consentire un ricambio equilibrato degli organi societari e l'elaborazione da parte delle società di idonee politiche per la selezione dei candidati, di qualsiasi sesso essi siano, dotati dei necessari requisiti di professionalità e competenza. Quando si concluderà il successivo *iter* parlamentare e il disegno di legge diventerà legge, l'Italia si porrà all'avanguardia in Europa, avendo anticipato le nuove misure legislative che, sul tema, ha già annunciato la Commissione europea. Concludo, ringraziando ancora il vice presidente della Commissione, senatore Ferrara, la relatrice e tutti i senatori e le senatrici. Governo, maggioranza e opposizione hanno avuto un confronto leale e proficuo ed è davvero gratificante poter dire di avere preso parte a un dibattito di così alto profilo.

Presidente, colleghi, la presenza delle donne nelle istituzioni e nei livelli decisionali è una conquista relativamente recente ed esigua. Purtroppo, consentitemi di aggiungere, quelle conquiste e quei passi avanti nell'emancipazione femminile che ci sembravano solo qualche anno fa procedere speditamente sembrano oggi segnare il passo, se non essersi fermati del tutto. La Costituzione italiana sancisce la parità tra uomo e donna attraverso il principio di eguaglianza, formale e sostanziale, previsto all'articolo 3, e stabilisce che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che (...) impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti (...) all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Sempre nell'ambito della Costituzione, l'articolo 51, primo «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge». L'8 marzo del 2003, su iniziativa della Commissione pari opportunità operante presso la Presidenza del Consiglio, all'articolo 51, primo comma, è stato aggiunto un secondo periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». In Europa, dove la parità tra donne e uomini è un diritto fondamentale e uno dei principi comuni dell'Unione europea, leggi per riequilibrare la presenza femminile nei consigli d'amministrazione delle aziende quotate in Borsa sono state già approvate in Norvegia, Islanda, Spagna e Francia, mentre sono al vaglio in Germania, Gran Bretagna, Austria e Belgio. L'Unione europea ha contribuito in maniera rilevante alla promozione della condizione femminile e al miglioramento della vita di donne e uomini elaborando molte norme sulla parità di trattamento tuttavia, nonostante l'evoluzione positiva verso una società e un mercato del lavoro più egualitari, le disparità tra donne e uomini persistono, principalmente a scapito delle prime. La vice presidente della Commissione europea e commissario per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, Viviane Reding, l'8 marzo scorso ha dichiarato che, se entro un anno le imprese europee non avranno fatto progressi per accrescere la partecipazione delle donne ai processi decisionali, saranno i legislatori europei ad intervenire con quote giuridicamente vincolanti, visto che l'obiettivo stabilito dall'Unione europea per i 27 Paesi aderenti

Nell'ultimo rapporto sull'uguaglianza di genere dell'Unione europea viene evidenziato che le aziende nei cui consigli di amministrazione è maggiore la presenza femminile hanno registrato *performance* migliori rispetto a quelle con CDA prevalentemente maschili. Alle stesse conclusioni è arrivato, in Italia, uno studio del Cerved Group per «CorrierEconomia» che ha svolto, nel triennio di attività 2007-2010, un'analisi sulle 2.000 maggiori aziende italiane (quelle che hanno fatturato oltre 100 milioni di euro nel 2008 o nel 2009). Dal suddetto studio è emerso che le imprese ai cui vertici c'è un numero maggiore di donne hanno conseguito risultati migliori, in maniera stabile, in tutti e tre gli anni analizzati. Infatti, i coefficienti che indicano la redditività e l'efficienza economica della gestione sono percentualmente più alti nelle aziende a maggior presenza femminile. Lo stesso è emerso, per quel che riguarda i problemi di insolvenza, il cui tasso di rischio non solo scende in presenza di un numero maggiore di donne, ma addirittura si dimezza quando c'è un presidente o un amministratore delegato donna.

Grazie, signor Presidente. Purtroppo, secondo lo stesso studio, nello stesso triennio 2007-2010, il bassissimo dato di imprese che vedono la presenza del 30 per cento di donne ai vertici è rimasto invariato intorno al 12 come invariato è rimasto il loro peso tra gli amministratori, solo il 9 per cento. Quindi, a fronte di una maggiore consapevolezza e riconoscimento del valore dell'impegno femminile, non vi è una corrispondente crescita della presenza del genere femminile nel mondo delle imprese. Inoltre, i risultati di uno studio promosso dalla Scuola di direzione aziendale dell'Università Bocconi, del settembre 2010, rivelano che, sul totale dei componenti degli organi sociali di 274 società quotate, soltanto il 7,6 per cento è di sesso femminile, con un lieve incremento rispetto ai dati del 2009 (in cui la percentuale era pari al 6,9 Il Consiglio d'Europa, in una raccomandazione del marzo 2003, ha sottolineato che una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nei processi decisionali è un'esigenza di mera giustizia e che «la parità dei sessi è elemento costitutivo, non negoziabile, della democrazia». È, quindi, nell'interesse della salute della nostra democrazia che bisogna raggiungere una parità effettiva sia nelle istituzioni che nella società, perché non è pensabile che la parte più numerosa dei cittadini italiani non sia adeguatamente presente in tutte le sedi in cui vengono prese decisioni per il funzionamento del nostro Paese. Allora che fare? Le cosiddette quote rosa si sono rivelate l'unico strumento efficace per non perdere i talenti femminili che esistono, ma che vengono solitamente esclusi dai ruoli decisionali. Le quote rosa, termine che noi donne per prime non amiamo (infatti, negli altri Paesi europei sono chiamate quote di genere), rappresentano un mezzo verso la parità di risultato: un mezzo tramite il quale sperare di poter realizzare un progetto

In questa prospettiva, le quote non devono essere una discriminazione nei confronti degli uomini, ma piuttosto una compensazione per le barriere strutturali che le donne incontrano nel processo elettivo. Non sussiste, più a mio parere, alcuna giustificazione del ritardo, come emerge dagli studi citati, considerato l'elevato livello di preparazione raggiunto dalle donne, in particolare nel campo dell'economia e della finanza, e quindi tale situazione richiede una riforma radicale del sistema, anche a livello culturale. In questa ottica, quindi, il provvedimento che stiamo per approvare costituisce il doveroso adempimento dell'obbligo previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 51 della nostra Carta costituzionale e una tappa fondamentale di un percorso importante per superare quelle barriere culturali che ancora oppongono resistenza all'emancipazione femminile e fanno sì che la donna, soprattutto nel mondo del lavoro sia ancora fortemente discriminata sia per tasso di occupazione che per differenza salariale. L'augurio è, quindi, che questo provvedimento di sostegno ad una maggiore presenza delle donne nei livelli decisionali, contribuisca a fare da volano per ridurre il divario fra i sessi in tutti gli ambiti. Sono certa che la norma che stiamo approvando sarà essenziale per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese perché contribuirà a garantire pari opportunità alle donne, ma anche ad incentivare la produttività aziendale. Infine, ci allineerà alle democrazie europee più avanzate e, per una volta, ci permetterà di essere in anticipo rispetto a quello che verrà presto chiesto dall'Unione europea, per la quale - cito dal rapporto della Commissione - «La parità di genere non è solo una questione dì diversità e di equità sociale ma costituisce anche uno dei presupposti per il raggiungimento degli obiettivi di crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale». Vorrei esprimere la mia particolare soddisfazione per l'attribuzione alla CONSOB di un potere regolamentare e sanzionatorio, nel caso in cui non venga rispettato il criterio di riparto per garantire l'equilibrio di genere,

quindi con la massima urgenza a valutare la possibilità che il Ministro per le pari opportunità promuova l'adozione di un codice di autoregolamentazione con cui le società aderenti si impegnano a riservare al genere meno rappresentato la quota prevista

Gli obiettivi dell'Unione europea in materia di uguaglianza tra donne e uomini hanno lo scopo di assicurare le pari opportunità e l'uguaglianza di trattamento tra donne e uomini, nonché di lottare contro ogni discriminazione basata sul sesso. Più della metà degli elettori europei è costituita da elettrici, ed è un dato di fatto che negli ultimi anni è aumentata la partecipazione delle donne alla vita economica dei Paesi e anche dell'Italia. La presenza femminile nei settori produttivi ha costituito una straordinaria fonte di vitalità e di innovazione per l'Italia, dimostrando di essere capace di rinnovarsi e di competere sui mercati internazionali in numerosi campi. Tuttavia, viviamo in un sistema sociale e culturale che rende molto difficile, per una donna che non voglia rinunciare alla famiglia, fare carriera. Più si sale nella scala gerarchica e più è arduo conciliare la sfera individuale con quella professionale. Sulla donna ricadono sostanzialmente i compiti di cura, dei figli *in primis*, ma anche dei genitori anziani, e di conduzione della casa. Questa situazione si riflette sui percorsi di carriera delle donne e sulla qualità della loro vita. Le donne al vertice delle imprese italiane sono poche, molto meno della media europea. Questo è un fenomeno purtroppo noto a tutti e di cui da qualche tempo giustamente si è iniziato a discutere. I dati diffusi dal Cerved, la società che gestisce le banche dati per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, testimoniano un tessuto imprenditoriale femminile molto vivace e competitivo, che ha retto l'urto della crisi meglio di quello maschile e che ha indotto gli analisti economici a parlare di un vero e proprio «fattore D», cioè fattore donna. Il problema è che ancora oggi in alcune realtà lavorative la presenza delle donne tende a scarseggiare. Ciò è soprattutto evidente nei consigli di amministrazione delle società quotate in Borsa. Infatti, se prendiamo come esempio i consigli di amministrazione delle prime trecento società europee, di cui 23 sono società italiane, la situazione vede il nostro Paese in una posizione ancora peggiore. La European Professional Women Network, che ogni due anni fotografa i consigli di amministrazione delle trecento società maggiori in Europa, annovera l'Italia, insieme al Portogallo, tra i Paesi ritardatari nella promozione di pari opportunità ai vertici aziendali. All'interno delle 23 società italiane censite sono 375 i seggi di consiglio di amministrazione disponibili;

Ciò spiega il penultimo posto, su 17, occupato dal nostro Paese nella classifica relativa alla presenza femminile nei consigli di amministrazione delle grandi imprese europee. Proprio in virtù di tali dati e di molte altre statistiche fatte all'interno del settore societario nei vari CDA si è avvertita la necessità di sostenere questa legge che pone l'obiettivo di riequilibrare l'accesso alle cariche direttive delle sole società quotate in borsa che, come si evince dai dati riportati, sono quasi *off-limits* per le donne e ciò nonostante il fatto che esse operino su un mercato regolamentato e impieghino modelli di gestione manageriale basati sulla professionalità degli amministratori piuttosto che che sull'*affectio societatis* dei singoli partecipanti all'impresa, come accade invece per le società di persone e per molte società a responsabilità limitata, di solito piccole e a conduzione familiare. Il presente disegno di legge costituisce dunque il doveroso adempimento di un obbligo costituzionale. Le disposizioni in esso contenute hanno lo scopo di promuovere le pari opportunità di donne e uomini nell'ambito delle amministrazioni pubbliche dello Stato, delle società pubbliche e a capitale misto e delle società per azioni quotate in borsa. Per questo motivo ci sentiamo in dovere di suggerire un percorso nuovo di crescita professionale delle donne al fine di porle effettivamente in posizione di vertice, nel senso di massima responsabilità, all'interno della società, nella consapevolezza dell'importanza di premiare e valorizzare le risorse professionali a prescindere dal sesso. Sono convinta che la presenza femminile nella composizione dei consigli di amministrazione si saprà far valere e che avrà effetti positivi sulla gestione delle imprese, come li ha avuti naturalmente in questo momento di di grave crisi economica, e spero che nel 2011 ancora non si debba tornare indietro nel tempo a quando la parità dei diritti uomo-donna era solo un'utopia. Al giorno d'oggi dovrebbe essere, non dico obbligatoria, ma quasi scontata, soprattutto in un Paese civilizzato e all'avanguardia come il nostro, visto che l'Italia ha sempre dimostrato di essere all'altezza di molte situazioni spesso complesse.

Signor Presidente, gentili membri del Governo, onorevoli colleghi senatori, innanzitutto i doverosi ringraziamenti e complimenti a tutti coloro che in queste settimane hanno lavorato al miglioramento di un testo arrivato dalla Camera con alcuni elementi di criticità, che hanno dovuto essere affrontati con estrema attenzione. Non è stato facile in queste settimane in 6a Commissione affrontare un tema di questa delicatezza, con le sensibilità molto diverse, e spesso contrapposte, esistenti tra noi membri della Commissione. E mi devo complimentare con il vice presidente, senatore Ferrara, con la relatrice, senatrice Germontani, e con il sottosegretario Sonia Viale, che, nel pieno rispetto dei loro ruoli, sono riusciti a gestire magistralmente le varie situazioni che si sono venute a creare durante i lavori della Commissione. Voglio dichiarare da subito il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord, un voto dovuto alla convinzione che il testo di questo provvedimento «difficile» è stato notevolmente migliorato, ma vorrei anche che agli atti dei lavori di quest'Aula rimangano alcuni spunti di riflessione che sottolineino solo alcuni dei dubbi che hanno accompagnato e accompagnano tuttora l'approvazione di questo provvedimento. Cercherò di farlo senza facili demagogie, senza voler contrastare a tutti i costi una tendenza - passatemi il termine - alla beatificazione di un provvedimento sicuramente più facile da osannare che da contrastare per il timore di accuse di non politicamente corretto. Nel dettaglio, quindi, stiamo andando a dare il via libera a tre mandati per i rinnovi nei CDA delle società quotate, con una prima tornata prevista per l'anno prossimo, per il 2012, nei consigli di amministrazione il 20 per cento dei consiglieri dovranno essere donne, per arrivare poi, a regime, al 30 per cento a partire dal 2015, nel secondo rinnovo. Sono in molti a ritenere che il testo licenziato dalla Commissione finanze del Senato sia equilibrato e frutto di un giusto compromesso tra la necessità di assicurare una maggiore partecipazione femminile e i timori delle aziende. Vorrei però cogliere questa occasione per esprimere una mia perplessità. Nei consigli di amministrazione, così come - in linea di massima - in qualsiasi altro ambito, non vorrei che fosse più significativa l'appartenenza ad un genere (sia esso maschile o femminile) rispetto alla reale competenza e capacità della persona. Parità di candidati di sesso maschile e femminile e parità di competenza. I problemi iniziano con l'unione di questi due presupposti. Siamo veramente sicuri che sarebbero scelte sempre le persone più preparate? Non sarebbero forse altri gli interventi utili per garantire una progettualità, l'innovazione e lo sviluppo della nostra economia? Un conto sono provvedimenti come la concessione di incentivi creditizi o fiscali, la rimozione di eventuali ostacoli (quali le difficoltà legate all'iscrizione dei propri figli agli asili nido, alle scuole materne)

E proprio in materia di discriminazione nell'*iter* di questo provvedimento qualche dubbio è sorto: non nascondiamocelo. Mi riferisco al principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della Costituzione.

A tale proposito si è espresso anche il cosiddetto Gender Equality Act, il documento di eguaglianza di genere che è stato il principio ispiratore di notevoli mutamenti

sono stati capaci di promulgare nuove leggi sia in favore delle pari opportunità, che contro la discriminazione. Tra questi mutamenti non possiamo non ricordare l'*Equal Pay for Equal Work* ovvero parità di salario per lo stesso lavoro a prescindere dal sesso. La verità però è che temo che questo disegno di legge possa infine rivelarsi discriminante nei confronti delle donne proprio per il fatto che parte dal presupposto che tutte le donne siano bisognose a prescindere, che tutte siano in difficoltà e che tutte, in linea di massima, rientrino nella cosiddetta fascia debole.

È un dato sicuramente incontrovertibile che nel nostro Paese, quanto a presenza femminile nei vertici aziendali, siamo molto indietro rispetto alla media europea. Ma qual è il vero motivo di tale arretratezza? Non certo, o non solo, la discriminazione di genere: piuttosto, sono diversi altri campi in cui noi come legislatori dovremmo impegnarci ad intervenire per arrivare ad una vera e propria parità. In queste settimane di discussione ho sentito molti richiami al sistema produttivo, economico e sociale della Norvegia - come dicevo prima - e della Scandinavia, più in generale. In Norvegia dove - come è più volte stato ricordato - le quote rosa nei CDA esistono dal 2006, le donne *manager* vengono soprannominate «gonne dorate» «gonne dorate» perché guardate come raccomandate di Stato. Nessuno dice però che lì la femminilizzazione dei CDA non ha determinato un aumento dell'efficienza e che, anzi, si è visto che, potendo scegliere, gli stessi consigli norvegesi a forte presenza femminile nel 98 per cento dei casi nominano amministratori delegati degli uomini. Questo non perché gli uomini siano più preparati delle donne, assolutamente no, ma perché le aziende reputano vitale poter scegliere liberamente da chi farsi guidare.

che il sistema Paese è completamente diverso dal nostro. Ci sono altri orari di lavoro, c'è una situazione economica ed occupazionale completamente diversa e c'è persino, da parte delle stesse donne scandinave, una concezione molto diversa del rapporto con l'altro sesso. sesso. Non credo che creare un privilegio femminile per legge, perché di legge stiamo parlando, tanto che sono previste persino le sanzioni (e addirittura, voglio sottolinearlo, la decadenza Le donne, a mio avviso, non hanno bisogno di privilegi, ma al limite di diritti e della possibilità che questi vengano sempre rispettati. Non sono certo intervenuto oggi in quest'Aula per smentire il fatto che ancora oggi, all'alba del XXI secolo, le donne abbiano ancora difficoltà ad affermarsi nel mondo del lavoro rispetto agli uomini. Credo però che un modo per riuscire a fare realmente un passo in avanti in materia di pari opportunità non sia certo quello di andare ad imporre altre leggi nel settore privato: come invece lavorare per creare, o incentivare, uno Stato sociale molto più efficiente e protettivo, con servizi a misura sia di uomo sia di donna. Pensiamo soltanto agli orari di lavoro nelle aziende private e negli uffici pubblici. È qui che vanno praticati tutti quegli interventi che permettono ad una donna di esprimersi nelle sue molteplici qualità: moglie, mamma e lavoratrice. non posso che concludere questo mio intervento con una riflessione. Se io fossi una donna, mi sentirei profondamente umiliata nel sapere che sono stata nominata consigliere di amministrazione solo per rispetto ad una normativa che altrimenti sarebbe costata all'azienda

non volete essere scelte per le vostre capacità e per i vostri meriti? E non pensate che le vostre capacità e i vostri meriti possano andare ben oltre questo 30 per cento fissato per legge?

Ne ricordo solo alcuni, a parte il diritto di voto acquisito nel 1946. Se vogliamo risalire alla storia, la prima legge che ha consentito alla donna di affacciarsi sullo scenario pubblico è stata la legge Crispi del 1890, 1890, che ha consentito alle donne di entrare nei consigli di amministrazione delle Opere Pie, delle IPAB. Quella legge ha rotto un tabù che, letto con gli occhi di oggi, era davvero abissale:

dell'articolo 51 della Costituzione fino ad arrivare, nel 2006, al codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Ho fatto questo *excursus*, molto velocemente, solo per ricordare alcune tappe.

Questo processo di uguaglianza investe non solo e non tanto il nostro Paese, ma tutta l'Europa e, se vogliamo, va oltre i confini europei perché investe l'intero pianeta.

una vera ed effettiva uguaglianza tra uomo e donna, saremo in grado di istituire l'uguaglianza tra l'uomo e tutto il creato». Questo è un piccolo passo, ma che va in tale direzione. oggi in discussione prevede strumenti volti a garantire la parità di accesso negli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati (e non solo) e rappresenta un successo per il genere femminile, ma mi permetto di sottolineare che dovrebbe rappresentarlo anche per il genere maschile e per l'intero Paese. Non si può non notare che, ad oggi, la presenza delle donne nei vertici societari costituisce una triste rarità. Secondo statistiche accreditate della Commissione europea, l'Italia si colloca solo al ventinovesimo posto su 33 Paesi censiti in materia di lavoro delle donne, precedendo la Repubblica di Malta, Cipro, Lussemburgo e Portogallo. A livello mondiale, poi, si colloca addirittura al settantaquattresimo posto, subito prima del Gambia. Eppure a livello europeo, già da tempo è stato intrapreso un percorso finalizzato proprio a porre le donne al centro della vita economica. Ad esempio, la Norvegia è stato il primo Paese ad introdurre un meccanismo legislativo volto a garantire la presenza di quote femminili nei vertici delle società società quotate, sancendo l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2006, di riservare alle donne una parte dei posti nell'ambito dei consigli di amministrazione delle società quotate. L'esempio norvegese è stato seguìto ed emulato dall'Olanda e dalla Francia ed altri Paesi hanno adottato misure *ad hoc* sempre finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo. L'Italia, dal canto suo, solo ora

commentando alcuni percorsi avvenuti proprio qui, al Senato, voglio ricordare che in Italia, secondo l'ultimo rapporto dell'Associazione fra società per azioni,

Nonostante le donne posseggano un elevato livello di istruzione, conseguito in tempi minori e con risultati migliori, di fatto sono poche quelle che hanno la possibilità di sedere nei consigli di amministrazione.

da una riserva del 30 per cento dei membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle società quotate in favore del genere meno rappresentato; si prevedeva l'entrata in vigore entro il termine di sei mesi

dal punto di vista culturale lancia un segnale significativo, e spero che, al di là delle società quotate in borsa, le prime ad applicare queste norme siano le società partecipate

seguirla, poi, è quanto di meglio c'è per gli uomini». Noi, oggi, possiamo fare molto di più che pronunciare la parola uguaglianza: possiamo seguirla e dimostrare al Paese di essere in grado di viverla. Speriamo di approvare il disegno di

di legge, hanno invocato il principio di uguaglianza di cui alla prima parte dell'articolo 3 a sostegno di una inopportunità, se non addirittura di una lesione dei principi costituzionali, dell'introduzione che si fa con questo provvedimento di una discriminazione positiva in favore delle donne per il loro ingresso nei CDA delle società quotate. I senatori e le senatrici, ma mi piace citare i senatori per primi, che hanno lavorato invece alla redazione di questo testo - e l'hanno fatto sia alla Camera che al Senato - sono consapevoli che l'introduzione di una discriminazione positiva, o di una quota per meglio definirla, secondo l'accezione comune, è esattamente integrativa, realizzatrice, attuativa di quella seconda parte dell'articolo 3 della Costituzione che allude appunto all'eguaglianza sostanziale.

le azioni positive rappresentano un movimento generale delle società avanzate; rappresentano, cioè, uno strumento della modernità che ha nella finalità dell'integrazione tra i sessi e nell'assunzione delle responsabilità collettive in sede politica, sociale ed economica uno dei pilastri per l'avanzamento delle società.

una discriminazione positiva: esse non sono altro, fuori da ogni furore ideologico, che uno strumento transitorio che serve ad accelerare un processo, che magari già è in atto, ma è in atto con modalità di una tale lentezza, e spesso di una tale scissione - e tornerò sull'argomento - da non riuscire a raggiungere il risultato che è quello, in questo caso, arricchire l'ambito dei soggetti ammessi alle opportunità economiche, dando così nuova prospettiva, ma direi nuova linfa e nuova propulsione, al settore economico e finanziario del Paese. di una norma transitoria. Ma perché parlavo di una società scissa? Perché credo che nessun collega in quest'Aula, qualunque sia il voto che esprimerà su questo testo, possa negare che oggi registriamo una scissione evidente: da un lato, infatti, le donne italiane hanno raggiunto, non solo nel campo dell'istruzione, ma anche nel campo dell'accesso alle professioni, e anche impieghi pubblici tra i più prestigiosi, una percentuale altissima; dall'altro, continuano a restare escluse dalle sedi delle decisioni, cioè esattamente quelle nelle quali questo aumento del talento, delle competenze, delle professionalità potrebbe essere un ulteriore motore per l'Italia che vuole crescere. Quello che abbiamo davanti è uno strumento che nasce negli Stati Uniti d'America - lo sappiamo tutti - e nasce esattamente per accelerare quel processo di integrazione che era stato aperto dalle grandi battaglie degli anni Sessanta e viene poi applicato anche a soggetti diversi, in questo caso alle donne. Si è detto in quest'Aula - secondo me adoperando un argomento non proprio, non efficace (in qualche modo lo diceva anche poc'anzi il collega Mura) - che il sistema delle quote è mortificativo del merito. del merito. Siccome le donne italiane sul merito hanno investito - almeno le ultime generazioni, e con risultati più che fruttuosi probabilmente bisognerebbe, colleghi, porsi un'altra domanda: non è che magari è esattamente il contrario, cioè che se non ci sono quote non ci sono occasioni per mostrare il merito e metterlo al servizio del Paese? E questo non è un problema delle donne italiane, ma delle classi dirigenti italiane, e se qui oggi molti senatori - io mi auguro la stragrande maggioranza, uomini e donne si esprimeranno in questo senso lo faranno esattamente perché, da classi dirigenti, si sono posti il problema di come dare nuova linfa, nuovo impulso e nuova ricchezza allo sviluppo dell'Italia. Certo, dà disturbo; certo, può probabilmente irritare: ma è esattamente il risultato che dobbiamo ottenere, quello di operare una rottura nei meccanismi che sempre replicano la medesima forma di esclusione, per torpidezza, per assuefazione e anche, lasciatemelo dire, colleghi, per convenienza. Il collega Mura dice: «se io fossi una donna(...)». Lei non è una donna, collega Mura! E alle moltissime ragazze che mi auguro ci stiano ascoltando piacerebbe essere, da donne, laureate, specializzate, professionalizzate, nelle stesse identiche condizioni di facilità di accesso e di opportunità per far valere il proprio merito che oggi sono riservate agli uomini. *(Applausi dal Ma io credo che ci sia da sottolineare anche un altro aspetto. Questa proposta nasce sia alla Camera che al Senato. Viene discussa per la prima volta

da voler dare un nome a questa legge, probabilmente sarebbe lunghissimo l'elenco dei nomi che dovrei mettere, tutti identicamente, in ordine alfabetico, sulla stessa riga: ci sarebbero donne, e anche degli uomini. Ma questo non è un fatto strano. Se noi rileggiamo la storia d'Italia degli ultimi anni possiamo vedere come

svolto tante deputate del centrosinistra, a cominciare da Elena Montecchi, ma che è stato poi assunto da Stefania Prestigiacomo. Io stessa che per la prima volta ho ricoperto il ruolo di Ministro per le pari opportunità ho visto molti miei

sono state capaci di tessere anche storie politiche molto diverse: certo, anche tra frizioni, debolezze, difficoltà, ma, normalmente, il risultato ottenuto è stato importante per l'Italia. ultime due questioni. In questa occasione - mi fa piacere dirlo davanti alla sottosegretaria Viale, che ha seguito con attenzione i nostri lavori e che io ringrazio anche per le parole che ha pronunciato in quest'Aula

che erano rimasti un po' spiazzati dalla definitività del provvedimento approvato dalla Camera. Io

che non sempre si vedano le donne italiane come sono, e per non vedere 200.000 professionisti in realtà ci vuole una lente assai opaca. Però credo che in questo ramo del Parlamento ci si è assunti ancora una volta una

ha lavorato, ed anche delle colleghe degli altri Gruppi parlamentari. È anche grazie alla loro determinazione, alla loro capacità di confronto e alla loro straordinaria autonomia - straordinaria lo aggiungo io, forse anche da avversaria politica - che questo risultato oggi si è raggiunto.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunge oggi in Aula un provvedimento che ha aperto un profondo dibattito all'interno dei sistemi economici e, più in generale, nel Paese. Un dibattito salutare che ha permesso innanzi tutto una nuova e aggiornata valutazione sui numeri della recente avanzata delle donne negli ambiti professionali e industriali, che negli ultimi venti anni ha cambiato il volto della nostra economia. L'articolo 3 della Costituzione afferma: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini,

È evidente la stringente connessione con l'articolo 41 della Costituzione, che garantisce la libertà dell'iniziativa economica privata, affermando al secondo

"La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". La normativa chiude il cerchio della promozione delle pari opportunità e della stagione delle azioni positive che irruppero nel dibattito parlamentare verso la fine degli anni Ottanta. In più di venti anni quelle azioni positive hanno prodotto risultati significativi nel sistema formativo e nelle professioni, poiché oggi le donne sono il 60 per cento dei laureati, il 42 per cento dei magistrati e degli avvocati, il 32 per cento cento degli imprenditori, il 12 per cento degli amministratori delegati e il 22 per cento dei *manager*. Siamo ancora ben lontani dal 60 per cento di partecipazione femminile al mercato del lavoro che ci indica l'Agenda di Lisbona;

Il dibattito su questi temi è ancora aperto, e non sarà l'approvazione della legge che probabilmente lo chiuderà. Esponenti del mondo economico e accademico ritengono che il sistema delle quote non rappresenti lo strumento migliore e più adatto a favorire la piena realizzazione di un riequilibrio tra i generi, così come anche senatori dei più diversi Gruppi non ritengono soddisfacenti i miglioramenti introdotti dalla Commissione finanze, che pure sono stati importanti e significativi, soprattutto in ordine alla costituzionalità e al permanere della decadenza dell'intero consiglio di amministrazione in caso di non ottemperanza della legge. Qualcuno arriva perfino a paventare il rischio di un potenziale scoraggiamento alle quotazioni in borsa che, al contrario, vanno favorite con misure non rigide. Ma il provvedimento sulle cosiddette quote rosa si inserisce nella tradizione della civiltà giuridica italiana, che ha sempre posto al centro della sua attenzione la tutela e la promozione della condizione femminile, assecondandone nel tempo la configurazione sociale. Vi è una contiguità che lega la legislazione a protezione della maternità del 1971 - una legge tuttora tra le più avanzate del mondo con altre norme che sono state approvate negli anni Settanta contro le discriminazioni in ragione del sesso sui luoghi di lavoro. E poi, come non ricordare la fondamentale legge generale per la realizzazione della parità professionale tra uomo e donna del 1991? Quella importante riforma, similmente a quanto accade oggi con le quote rose, non si limitò a recepire sul piano normativo i risultati di una già avvenuta e realizzata evoluzione sociale ed organizzativa, ma anticipò e orientò, per indirizzarlo e guidarlo, il cambiamento verso una cultura di gestione delle imprese private, ma anche degli enti pubblici, che valorizzasse una loro complessiva qualità competitiva attraverso la valorizzazione della specificità femminile. Per la prima volta entrò nell'esperienza giuridica italiana la nozione delle azioni positive come quotidiano strumento organizzativo, per rendere concreta, e dunque vera, la realizzazione del principio di uguaglianza. Nella stessa scia si colloca questo provvedimento a cui il Popolo della Libertà ha dato un contribuito positivo sia nel suo avvio nella discussione alla Camera dei deputati, sia nel suo migliore arricchimento di contenuti nel lavoro fatto in Commissione qui al Senato. È stato un lavoro serio quello compiuto a Palazzo Madama con il positivo contributo di tutti, anche per rendere più italiano, e cioè più efficace e penetrante, il meccanismo giuridico dell'intervento di promozione della rappresentanza femminile nei luoghi di decisione e di comando delle grandi imprese nazionali. Sono stati infatti superati alcuni aspetti che non avrebbero favorito, con la loro rigidità, il pieno dispiegamento degli effetti della normativa, il quale può essere garantito solo dalla conciliazione consapevole tra le istanze etiche e quelle organizzative, tra la tutela dei diritti e la tutela delle precondizioni economiche che rendono i diritti effettivamente esigibili. In questo senso, il disegno di legge, così come migliorato, allinea la legislazione italiana ai migliori standard europei. Come ogni azione positiva degna del suo nome, quella introdotta da questa legge ha natura straordinaria e dunque limitata nel tempo, e i suoi effetti, cari colleghi, dovranno essere monitorati e verificati sul campo. Lo dico con grande franchezza, consapevole dell'appassionato e serrato dibattito che c'è stato e anche delle opinioni diverse che, legittimamente, sono emerse. Dovremo accuratamente vigilare affinché, per esempio, nei consigli di amministrazione entrino donne dal forte talento manageriale, con un effetto virtuoso di trazione su tutto il *management* femminile, e non presenze di comodo volte solo ad ottemperare agli obblighi della legge. Dovremo evitare che la normativa adottata si traduca, contraddicendo lo spirito di libertà e di favore all'intrapresa che il Governo ha dichiarato di voler mettere in circolo con la riforma la riforma dell'articolo 41 della Costituzione, in un appesantimento burocratico alla funzionalità degli organi di governo delle aziende maggiori. Dovremo fare in modo che le società più complesse, contrassegnate da assetti proprietari organizzati in maggioranze e minoranze strutturate e regolate da sofisticati patti di sindacato, non vengano paralizzate nelle dinamiche gestionali. Dovremo insomma evitare un doppio mercato, come avvenuto, per l'effetto di alcune leggi, tra le piccole imprese, più flessibili, più dinamiche, meno vincolate, e le grandi imprese, più irrigidite. Sarà quindi una sfida importante la verifica sul campo. Guai se le imprese medie a vocazione internazionale, che sono il cuore pulsante del nostro sviluppo, rinunziassero alla borsa per evitare i rischi di quote, e guai se le grandi imprese ritenessero conveniente allocare altrove i loro centri direzionali. Se sapremo coniugare maturità civile e dinamicità gestionale, valorizzazione delle competenze femminili e competitività delle imprese, controllo legale e libertà organizzativa, avremo compiuto un passo decisivo per vincere la grande sfida della modernizzazione italiana. Il riequilibrio del rapporto all'interno della società, della pubblica amministrazione, del mondo dell'economia e della politica deve essere soprattutto, però, frutto di un'azione volontaria. Quando ebbi la responsabilità di un Ministero, mi proposi, senza alcun vincolo di legge che me lo imponesse, di nominare una maggioranza di donne tra i direttori generali.

ringraziare tutti i componenti del Popolo delle Libertà in Commissione finanze, il vice presidente Ferrara, il capogruppo Conti, la senatrice Bonfrisco, tutti i colleghi di tutti i Gruppi che hanno contribuito ad elaborare il testo che arriva oggi dalla sede redigente, nonché la relatrice. Il Popolo della Libertà auspica che una scelta così forte aiuti tutti i protagonisti,

seconda: per rispettare l'opinione diversa di chi volesse esprimerla, perché la libertà, la democrazia e l'attività legislativa sono anche questo. Grazie, signor Presidente. Grazie ai colleghi che hanno portato a termine questa impresa. Grazie, soprattutto, alle donne, che contribuiranno al miglior governo della nostra economia del futuro.

perché continuerò a dire quello che ho detto fin dagli anni Ottanta, cioè da quando, nel 1983, ho iniziato la mia carriera politica, quando snocciolavamo ancora più o meno le stesse percentuali, quando incominciavamo a parlare delle quote e quando probabilmente poteva forse avere anche un senso parlare di quote, visto che si tratta di non è certamente così, perché parlarne ancora adesso, perdonatemi, significa riconoscere il fallimento non soltanto del Parlamento, ma di un'intera società che non è riuscita a creare una cultura diffusa

Non mi aspettavo l'applauso, perché mi sembrava ci fosse una convergenza su questo. Naturalmente desidero rivolgere il mio apprezzamento totale alle donne che, invece, credono nel discorso delle quote e hanno svolto con impegno e dignità il loro lavoro in in Parlamento perché evidentemente, a fronte di un fallimento, hanno ritenuto che oggi, sia pure nel terzo millennio, il tema delle quote continua ad essere di attualità e rispetto al quale c'è una sorta di necessità - non voglio parlare di urgenza, dopo tanti

un anno o un terzo appeso tra due anni e che poi ci sia la gradualità. Non credo che Nilde Iotti sia stata Presidente della Camera in quota; non credo che la Marcegaglia sia presidente di Confindustria in quota. Francamente non ci credo proprio. Posso pensare che probabilmente abbiamo maggiori difficoltà, che non sia stata data adeguata attenzione al tema, per esempio, del *welfare*, dei servizi sociali, della politica di conciliazione, della politica della famiglia e su tutta una serie di interventi dei quali parliamo ormai da tanti anni, ma rispetto ai quali non siamo riusciti a fare nulla o quasi, tant'è che oggi, a distanza di tanti anni, ancora snoccioliamo le nostri percentuali e ancora siamo ridotti a giocare di rimessa per tentare di fare in modo che ci sia qualcuno che voglia prendere in considerazione le professionalità femminili.

credo che ancora una volta mi troverò d'accordo con la collega Bonino, con la quale ho amichevolmente scambiato qualche idea poco fa. Per evitare d'esprimere un voto, sia pure di astensione, m'asterrò dal votare in modo tale che quest'Aula possa comunque conseguire la sua unanimità.

Entro stasera il Senato è chiamato a deliberare sulla costituzione in giudizio su un conflitto di attribuzione sollevato dalla corte d'appello di Roma, il cui deposito della memoria scade domani. È evidente che va deliberato in serata.

proprio per la sua solennità, e anche per consentire a chi non la pensava in un certo modo di dirlo. Di tutto mi si potrà accusare tranne che di non aver garantito proprio la libertà di espressione in Aula.

sarò costretto nel caso di sforamenti - vi chiedo scusa in anticipo - a togliere i tempi per rispettare anche il calendario dei lavori, che vede la deliberazione della costituzione in giudizio, il cui termine scade domani. Altrimenti, sarei sicuramente più generoso. Vi ringrazio in anticipo per la vostra comprensione. onorevoli colleghi, ho seguito con estremo rispetto il lavoro che ha accompagnato la discussione di questo disegno di legge fino all'attuale compromesso che state per approvare. D'altronde, il dibattito sulle quote ha caratterizzato tutto il movimento femminile nel nostro Paese. Mi auguro che abbiate ragione voi. Eppure non mi sono convinta, per ragioni di metodo e di merito. Di metodo: non condivido e mi sforzo di non praticare una politica per la quale il fine giustifica i mezzi. PdL).* Per favore! Non mi applaudite mai, normalmente. Se potete evitare anche oggi degli applausi un po' interessati, quando non "pelosi", ve ne sarei grata. Anzi, sono sempre più convinta che i mezzi prefigurano i fini, sicché non voglio arrendermi a considerare positivo il mezzo e il fine di una società organizzata per quote: tot bianchi e tot neri, tot uomini e tot donne, tot immmigrati, tot autoctoni, tot del Sud e tot del Nord, tot giovani e tot vecchi. Ma continuo a lavorare per una società basata sull'individuo e sul merito: criterio spesso invocato, quasi mai praticato, e in assenza del quale non è difficile prevedere da quali filiere familiari, elettorali, per non dire clientelari si tenderà a scegliere o meglio cooptare le componenti di queste quote. Legalizzarlo non aiuta. So perfettamente che molte amiche con cui ho lavorato, e con cui spero di continuare a lavorare, per la valorizzazione del patrimonio al femminile del nostro Paese sono entusiaste di questa misura. Altre, l'accettano quasi per sfinimento, per rassegnazione, vista la situazione davvero patetica in cui versano le bravissime donne italiane presenti in tutti i settori della società, ma impedite ad accedere ai ruoli decisionali, a partire, ovviamente, da quelli politici.

i limiti temporali previsti in questo disegno di legge, per i limiti del campo di applicazione. Perché mai sono escluse le società pubbliche? E, soprattutto, perché il temporaneo, nel sistema italiano, si traduce in permanente. Continuo a pensare in modo Continuo a pensare in modo più proficuo, e spero che lo faremo insieme, per lavorare per l'istituzione di un'Autorità indipendente contro le discriminazioni di genere, come vuole la direttiva europea, contro gli stereotipi limitanti, quando non umilianti, e perché i risparmi provenienti dall'equiparazione dell'età pensionabile siano utilizzati finalmente per una politica attiva che sollevi le donne italiane da quei servizi di assistenza e cura dei bambini e degli anziani che ad oggi gravano esclusivamente su di loro. Per questo noi tre radicali non parteciperemo al voto, ma spero che la differenza di oggi non ostacoli un lavoro comune su quelle altre politiche di cui siamo tutte quante appassionate.

Mi limito a dire una sola cosa: credo che il testo sia in più parti assolutamente faticoso e non condivisibile, ma non è tuttavia questa la ragione per cui ho deciso di chiamarmi fuori della sua approvazione. La ragione invece è che questa legge, voluta e fortemente sostenuta dalle colleghe senatrici in questa Camera (da donne cioè di cui ho non condizionata stima e considerazione, con cui peraltro condivido il privilegio di poter essere parte della massima istituzione del mio Paese), istituzione del mio Paese), è, a mio modo di vedere, inescusabilmente ingiuriosa nei confronti di quelle altre donne che, in alcuni casi essendo maggioranza, svolgono la funzione di magistrato, la professione di notaio, di avvocato, di medico, di ingegnere, di quant'altro, nella quotidianità, segnando i risultati del loro lavoro senza differenza alcuna rispetto a quegli uomini che svolgono le stesse attività. Sono donne che tutto ciò fanno, per aver superato esami, per aver affrontato concorsi, per essersi misurate alla pari. Sono donne che non hanno avuto bisogno, che non hanno chiesto, che non hanno ottenuto alcuna scorciatoia, alcun privilegio, alcun vantaggio. Ho viaggiato la scorsa settimana su un aeroplano comandato da una donna, non bella e non brutta (tanto per prevenire stereotipi di giornata), che - quando ha spinto i comandi perché fossero raggiunte le velocità che tutti conosciamo - non l'ha fatto per legge o per quota. Né in forza di una qualsivoglia scorciatoia, come questa legge in definitiva è. L'ha fatto semplicemente perché era capace. Se fosse uso dare un titolo agli interventi in Aula, non mi priverei, per questo mio di oggi, del gusto della battuta, dunque lo chiamerei senz'altro "donne che odiano altre donne". Ma poiché non ho la minima intenzione di praticare un tale esercizio, nemmeno per battuta, comunico che, in dissenso dal mio Gruppo, pur restando ovviamente presente in Aula, non prenderò parte alla votazione, e quindi non voterò il disegno di legge. [**VOTAZIONI QUALIFICATE Signor Presidente, trovo che la normativa in merito alle quote rosa sia sbagliata. Capisco e condivido le intenzioni di partenza che hanno spinto verso questa legge, ossia aumentare la presenza femminile nei luoghi che contano, quali i consigli di amministrazione delle aziende, ma mi chiedo se l'obbligatorietà per legge sia la soluzione migliore. Personalmente penso di no, e dubito che lo Stato possa interferire a tal punto. Trovo questa decisione profondamente sbagliata: non deve essere il sesso di una persona il criterio determinante e qualificante per il suo ingresso all'interno di un consiglio di amministrazione Si deve valutare quella persona per le sue capacità e competenze professionali e, se serve, per le sue doti personali: sulla base di queste valutazioni si può decidere per il sì o per il no, ma di certo non può essere il sesso della persona il metro di valutazione. Un sistema delle quote rosa così pensato è lontano dal mondo reale e dalla sua essenza, assolutamente contrario al principio di meritocrazia e lesivo nei confronti di quanti hanno competenza e capacità per ricoprire un determinato incarico. Un sistema siffatto equivale a valorizzare e premiare qualcuno non per quello che vale e per i suoi meriti, ma per la sua appartenenza ad un genere, a una minoranza, a un'etnia o ad una religione. Il principio in astratto può anche essere corretto, ma nella sua applicazione diventa iniquo. Nella gestione di un'azienda o della cosa pubblica devono prevalere ben altri principi e criteri, soprattutto quelli del merito e delle capacità individuali di una persona. Non credo che sia giusto distinguere tra uomini e donne, ma tra persone capaci e persone incapaci per ricoprire uno specifico ruolo e se ci sono capaci sia tra gli uomini che tra le donne, senza dubbio.

Chiunque si sia impegnato a favore della tutela e della promozione delle pari opportunità sa che in tanto le azioni positive sono efficaci in quanto siano coerenti con il contesto culturale e organizzativo nel quale devono andare ad incidere. Questo disegno di legge segue una strada diversa: una strada astratta, ideologica, e dunque giacobina. Sarebbe stato molto meglio estendere ed espandere la nozione di discriminazione indiretta prevista dall'articolo 4 della legge n. 125 del 1991 sino a ricomprendervi i casi in cui non ci sia corrispondenza

non c'è dubbio che il testo pervenutoci dalla Camera sia stato profondamente modificato e, a mio giudizio, migliorato in Commissione finanze.

un po' meno giacobini, se posso citare l'espressione del senatore Castro. Riconosciuti questi meriti, anche con i colleghi della Commissione finanze, resta in me un certo disagio nell'aver avvertito proprio nelle ultime giornate del lavoro in Commissione un

quasi intimidito rispetto all'orientamento della Commissione. È comprensibile, ma siccome mi auguro che così non sia né appaia alla Camera,

Signor Presidente, non nascondo l'imbarazzo, perché è la prima volta in quattro legislature che annuncio un voto contrario quando il mio Capogruppo invece si è espresso diversamente: lo faccio perché sono profondamente convinto che sia una legge inopportuna, inidonea allo scopo e assolutamente illegittima.

ma ricordo che un grande principio sostenuto da Einaudi era quello dell'uguaglianza dei punti di partenza, cioè della parità delle opportunità, non dell'uguaglianza dei punti di arrivo e della garanzia dei risultati. Questa formula, cari colleghi, è tradotta in maniera esemplare nella nostra Costituzione, che nei suoi articoli recepisce questo grande principio liberale. All'articolo 3, secondo comma,

della Costituzione, di rimozione di ostacoli e, all'articolo 51, novellato nel 2003, di pari opportunità, non di pari risultati e di pari mete raggiunte.

nei consigli comunali, nei consigli provinciali, o nei consigli regionali di una quota minima di uomini e di donne: è la stessa cosa, la stessa logica, lo stesso principio.

tradendo un principio sacrosanto sancito dalla nostra Costituzione in un campo delicato, quale quello della borsa, che coniuga l'impresa e il risparmio, l'industria e la finanza; finanza; prevede poi sanzioni gravissime per chi non ottemperi alla norma, fino ad arrivare alla decadenza; include i collegi sindacali, che non hanno nulla a che vedere con le problematiche espresse dai colleghi e dalle colleghe sostenitori della legge e, infine, stabilisce un regime particolare

Ministro delle pari opportunità cancellando il termine «parità di accesso tra donne e uomini» e tornando al concetto di pari opportunità. In sostanza, la scelta del Governo, avallata poi dal Parlamento, fu quella di confermare quanto hanno scritto peraltro autorevolmente anche Ruffolo e Baldassarre), riportando il testo della Corte costituzionale, secondo cui le finalità indicate dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione si propongono di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, non di attribuire loro direttamente quei risultati. In questo modo, nel 1995, la Corte cancellò la legge del 1994 relativamente all'alternanza uomo/donna nel proporzionale perché, scrisse:

chi paga quando poi, se non ottempera, nello stesso consiglio si vede decaduto. Avrei anche potuto votare a favore di questa legge - e questa era anche opinione del Governo, considerati gli emendamenti presentati in Commissione - se ci si fosse limitati alla diffida e alla sanzione pecuniaria.

relativo alla decadenza del consiglio di amministrazione. Concludo affermando che, anche se la norma è presentata come transitoria, si tratta di sospendere

Sono certo che ci saranno occasioni in Parlamento per discutere di provvedimenti tesi a rimuovere gli ostacoli, come dice la Costituzione, che impediscono la piena espressione e quindi il riconoscimento della piena parità, delle pari *chances* e delle pari opportunità. Questo provvedimento rimane nella logica delle quote, sistema elaborato ed attuato in ogni ordinamento per la tutela di categorie da proteggere, definizione che non può attribuirsi ai cittadini di sesso femminile. Tale approccio elude il principio di uguaglianza di ogni cittadino senza discriminazioni di sesso, razza o religione. Ma ciò che è più grave è che questo approccio ci allontana dalla necessità di lavorare per la modifica di un sistema economico e di un sistema politico costruiti, questi sì, su un modello maschile di organizzazione, che, non riconoscendo differenze nelle esigenze e nelle aspettative di piena realizzazione, discrimina e continuerà a discriminare nelle *chances* e nelle opportunità.

citate dall'autorevole collega Poli Bortone, per il fatto che a nessun loro collega, dipendente comunale, cittadino, verrà mai in mente che ricoprono ruoli chiave dell'amministrazione in quanto donne. Presidente, sono molto favorevole ad una forte presenza di donne negli organi decisionali. Quando ne ho avuto modo, le ho votate in moltissime occasioni, forse nella maggior parte. Ma vorrei continuare a scegliere, o ad essere scelto, a considerare le persone, o ad essere considerato, non in base al sesso o ad altre sorpassate e dannose divisioni nella società, ma in base alle idee e al merito: criterio che l'Italia avrebbe estremo bisogno di potenziare, ma che oggi farà un passo indietro. Per questo, con rispetto per il lavoro svolto da tanti stimati colleghe e colleghi, che ha migliorato il testo licenziato dal ramo più numeroso del Parlamento, mi asterrò.

*(PdL)*. Signor Presidente, signore e signori del Senato, in quest'Aula, pochi minuti fa, la senatrice Bonino ha mostrato fastidio per alcuni applausi che provenivano da queste file, compreso il mio, dicendo che respingeva gli applausi perché interessati.

io questa legge non la voto, e non la voto perché non mi piace, e se non mi piace non la voto. Non la voto perché il senso estetico, come dice il grande filosofo, è alla base della nostra scala di valori, non la voto perché amo molto le donne, ma soprattutto le rispetto molto di più di quanto le ami. E poi... l'ho promesso ad una mia amica.

Onorevoli colleghi, nella giornata di venerdì scorso un sisma di gravissima intensità ha colpito il Giappone, provocando migliaia di vittime. Pochi minuti dopo, una serie di onde anomale alte diversi metri si è abbattuta sulle coste seminando morte e distruzione. Le notizie che di ora in ora giungono dalle agenzie di stampa tracciano purtroppo un profilo sempre più grave dell'entità dei danni e del numero delle vittime e dei dispersi. Non appena appresa la notizia della devastante calamità che ha colpito il Giappone, ho espresso in un messaggio inviato al Presidente della Camera dei consiglieri, a nome dell'intero Senato, i sentimenti della più profonda solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita. L'assoluta gravità degli eventi che hanno colpito il popolo giapponese ha suscitato in tutto il mondo sentimenti di grande commozione. Il nostro Paese ha offerto immediatamente il proprio aiuto e la propria assistenza. Tutte le istituzioni nazionali ed europee sono chiamate ad una partecipazione senza riserve. Questo è un preciso dovere morale di fronte ad una catastrofe umana disarmante che ci lascia tutti sgomenti. In segno di cordoglio per le vite spezzate da questa immane tragedia e di vicinanza della nostra Istituzione alla sofferenza della popolazione giapponese, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

Con ricorso del 20 gennaio 2010, la Corte di appello di Roma -Sezione Prima civile - ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 30 giugno 2004 ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal senatore Roberto Castelli - oggetto di una vicenda processuale che ha come parte l'onorevole Oliviero Diliberto - costituivano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadevano, pertanto, nell'ipotesi di immunità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 7 febbraio 2011, n. 38, depositata in cancelleria il successivo 9 febbraio e notificata al Senato il 24 febbraio Nella seduta odierna la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso nel senso che il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto. Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Lega Nord voterà a favore della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità in ordine alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d'appello di Roma nel giugno 2010 e già dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale nell'udienza del 7 febbraio.

che ha riconosciuto insindacabile *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione la frase pronunciata dall'allora ministro della giustizia Castelli nel corso della trasmissione televisiva Quella frase è stata ritenuta nel 2004 dal Senato opinione espressa nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare e priva di ogni idoneità lesiva, se vista come espressione di un diritto di critica politica. Ricordo che per quella stessa frase pende anche un procedimento penale per diffamazione. Il Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nella sua relazione ha ricordato che si tratta della quinta occasione in cui la Giunta e l'Assemblea si trovano a dover affrontare la vicenda di quella frase resa nella trasmissione televisiva

Non dimentichiamo poi che il 22 luglio 2009, sempre per lo stesso caso, abbiamo adottato anche una deliberazione di diniego dell'autorizzazione a procedere per la ritenuta ministerialità del reato, sussistendo una delle finalità di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989. Riteniamo che questa deliberazione dell'Assemblea del Senato abbia natura sostanziale

Noi comunque voteremo a favore della proposta confidando in un ripensamento da parte della Corte costituzionale rispetto al suo orientamento restrittivo nell'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione Costituzione per accedere ad una nozione di nesso funzionale più conferente al mutato quadro socio-politico di riferimento e ritenendo dunque coperta dalla garanzia di insindacabilità qualunque attività riconducibile al mandato parlamentare.

nel saltellare canticchiando «Chi non salta italiano è». Io mi vergogno di dover votare un provvedimento offensivo del nostro Paese Il senatore Castelli si sente italiano quando vuole che i contribuenti italiani gli paghino un avvocato per il conflitto di attribuzione: si ricordi di essere italiano e rispetti il nostro Paese

da parte del senatore Castelli, fosse già oggetto di una delibera di questo Senato che è intervenuta nel luglio 2009; se fosse stato già deciso che il senatore Castelli, con quelle espressioni - lo dico solo per connotarle e per fare capire di che parliamo in quest'Aula perché poi se sono offensive al punto della diffamazione dovrebbe deciderlo un giudice

e che quindi stava difendendo le prerogative e l'esercizio della funzione di Governo nell'interesse supremo della Repubblica, come avete votato voi della maggioranza nel luglio 2009; se tutto questo fosse vero, il Senato non avrebbe ragione di sollevare con una sua delibera questa sera un conflitto di attribuzione in un ambito che è diverso da quello che vi ho ricordato e che ci ha ricordato il senatore Mazzatorta. La proposta che oggi ci perviene, approvata a maggioranza dalla Giunta, è di sostenere che le affermazioni del senatore Castelli sono insindacabili ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. Ebbene, vorrei ricordarvi che su questo stesso caso il Senato si è già espresso e ha sollevato un precedente conflitto di attribuzione.

ha dato torto al Senato dicendo, in maniera molto esplicita, che le dichiarazioni del senatore Castelli - le stesse che noi oggi abbiamo al nostro vaglio - non sono coperte da insindacabilità perché non sono legate a nessun atto né tipico né atipico compiuto nella funzione parlamentare e quindi la tutela dell'articolo 68, correttamente applicato secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, non opera. Questa sentenza non è di cento anni fa: è del luglio 2007. Quindi, la nostra prima attenzione come Senato dovrebbe essere quella di non riproporre alla Corte costituzionale che ci ha già dato torto

Quindi, essere bastonati - scusatemi l'espressione non parlamentare - due volte sulla stessa materia e sullo stesso fatto da parte della Corte costituzionale a mio modestissimo avviso, ma credo anche di molti colleghi del Partito Democratico che voterà no alla sollevazione del conflitto di attribuzione, è del tutto insensato, perché rappresenterebbe un'ostinazione masochistica nel farci dire dalla Corte costituzionale che non abbiamo capito come si applica l'articolo 68 della Costituzione.

si crede che l'articolo 68 copra le affermazioni fatte da un parlamentare non nell'esercizio della sua funzione parlamentare, ma perché fa politica e quindi fa politica dove e come vuole dicendo a sparlando come vuole.

caratterizza tutti gli altri cittadini italiani e che egli, oltre che a poter insultare (e insultarci) in quest'Aula, nelle relazioni che accompagnano i disegni di legge, nelle interrogazioni e in tutti gli atti collegati alla nostra attività parlamentare, lo può fare fuori di qui nei confronti degli altri cittadini. Questo oggi la nostra Costituzione non lo afferma e non ritengo utile cercare di farglielo dire a spese dello Stato, del contribuente, con difese tecniche onerose che vengono drammaticamente respinte dalle sentenze della Corte. Da ultimo, si dice: un Ministro parlamentare, che quindi non ha a disposizione sempre l'Aula, gli atti di sindacato ispettivo e non presenta individualmente

Ma dobbiamo aggiungere (oltre al rilievo che ho citato in apertura del mio intervento, che il Ministro di un Governo e il Presidente del Consiglio hanno un'altra disposizione costituzionale, l'articolo 96, che li protegge nell'esercizio della loro funzione)

siede tra i banchi del Governo, e quando vuol dire qualcosa che appartiene alla sua sfera d'espressione politica parlamentare sale sui banchi del PdL e le suona e le canta come le vuol dire e ottiene, per questo motivo, tutta la tutela parlamentare che ottiene il

nella qualità di Ministro della giustizia in carica. Dall'altra parte c'era un ex Ministro della giustizia. Ma non le viene il dubbio che una persona che ricopre il ruolo di Ministro della giustizia non possa ricorrere ad una forzatura dell'immunità parlamentare e debba, invece, per dovere civile e politico, presentarsi davanti ai giudici?

è l'ennesimo capitolo di una storia che ha avuto molteplici risvolti dal punto di vista giudiziario, ed ha visto il susseguirsi di una serie di giudizi e di pronunce, anche da parte della Corte costituzionale, ma, soprattutto, di numerose deliberazioni assunte da questa Assemblea in merito alla sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, in una fase iniziale e, successivamente, in in ordine dell'applicazione dell'articolo 96 della Costituzione, per la qualificazione ministeriale delle ipotesi di reato contestate al senatore Castelli. In linea con tutte le decisioni assunte, prima dalla Giunta e successivamente dall'Assemblea, oggi siamo qui a deliberare in ordine alla costituzione in giudizio del Senato in merito al ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte di appello di Roma nel giudizio civile che aveva visto il primo grado risolversi in senso favorevole - per così dire - alla posizione del senatore Castelli, poiché era stata accolta l'eccezione sulla non sindacabilità delle opinioni espresse, avendo il giudice di primo grado (il tribunale di Roma) ritenuto che le esternazioni di cui appunto il senatore Castelli era stato autore nel corso

Il conflitto di attribuzione promosso muove ovviamente da una lettura diversa della latitudine di protezione che offre la norma costituzionale, anche se temporalmente interviene quando quest'Assemblea - come è stato ricordato precedentemente - nel luglio del 2009 ha deliberato in ordine alla qualificazione come ministeriale delle ipotesi di reato relativamente al concorrente giudizio promosso in sede penale nei confronti del senatore Castelli. Ovviamente la qualificazione assunta dall'Assemblea del Senato può essere un elemento importante, di portata anche dirimente, rispetto alla decisione che dovrà essere assunta all'esito del giudizio civile. Il primo elemento per poter introdurre questo argomento nel giudizio civile è che il Senato si costituisca e possa in quella sede, attraverso l'utilizzo dei normali dei normali strumenti di difesa previsti nel giudizio per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, innanzitutto prospettare questo nuovo, successivo, ulteriore e, per molti versi assorbente, argomento. In ogni caso, la necessità della costituzione in giudizio risponde anche ad una prassi che il Senato ha sempre seguito. Mi permetto di dire, in dissenso pieno dalle considerazioni egregiamente svolte dal collega Sanna,

rappresenta l'occasione ulteriore per concorrere a definire in maniera puntuale quali sono i limiti dell'esercizio, nell'ambito delle funzioni parlamentari, del diritto di critica e la protezione più in generale della funzione parlamentare, la quale potrebbe ricevere una ricevere una protezione minore se tutte queste ragioni non venissero adeguatamente svolte e rappresentate nel corso del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.

della proposta rassegnata dalla Giunta in ordine alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d'appello di Roma.

come lei avrà potuto notare, in questa lunga vicenda non sono mai intervenuto perché ovviamente mi sono sempre rimesso all'Aula, e anche oggi non voterò. Questo è chiaro. Tuttavia, poiché il collega Sanna mi ha chiamato direttamente in causa,

credo sia giusto che i colleghi sappiano come essa è nata e come si è svolta. Dalla registrazione televisiva e dagli atti del processo l'onorevole Diliberto, di fronte ad una mia frase (sicuramente eccessiva, ma come in televisione se ne scambiano tantissime tutti giorni), mi disse testualmente: «Il mio partito ha bisogno di soldi. Ti querelo e ti faccio causa civile». Questa è l'alta motivazione per la quale l'onorevole Diliberto è andato avanti tutti questi anni. Mi sono offerto, anche attraverso i miei avvocati, di arrivare ad una transazione amichevole, perché ritengo che occupare un tribunale penale, un tribunale civile, il Parlamento e la Corte costituzionale

molto indegnamente - il Ministro. Questa è la pura verità dei fatti: ci sono gli atti processuali, ci sono le registrazioni, ci sono le testimonianze.

per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d'appello di Roma - Sezione Prima civile.

al fine di verificare la possibilità di giungere ad un atto di indirizzo unitario. Chiedo alla senatrice Bianconi se è stato definito un testo condiviso.

un testo unitario, al quale si riferiranno le dichiarazioni di voto. Credo che ciò rappresenti per il Parlamento una bellissima pagina di grande unitarietà

*(PD)*. Signor Presidente, anch'io voglio esprimere la grande soddisfazione del mio Gruppo per il risultato che siamo riuscite a ottenere stamani. Devo innanzitutto ringraziare le colleghe del mio Gruppo dell'opposizione, le colleghe della maggioranza e il Governo, nella persona della ministra Mara Carfagna, per il risultato che siamo riuscite a conseguire, che non era scontato in partenza. È il frutto di un lavoro comune: l'ordine del giorno è stato letteralmente scritto insieme. Naturalmente si è svolta una discussione a tratti vivace ed appassionata, nella comune consapevolezza della posizione in cui le donne si trovano nella rappresentazione che i *media* ne danno: tuttavia, siamo riuscite a trovare convergenze, sia nelle premesse che soprattutto nel dispositivo, che è risultato molto articolato e molto ricco.

Vorrei spiegare ai colleghi maschi appartenenti a tutti gli schieramenti il senso del nostro impegno affinché si trovassero punti di convergenza tra maggioranza, opposizione e Governo. Questo impegno, signor Presidente e colleghi, deriva da un convincimento profondo, per quanto mi riguarda. Quando si tratta del corpo delle donne, o quando si tratta di provvedimenti che mirano a far guadagnare potere alle donne - ne abbiamo discusso prima a proposito delle quote - la trasversalità costituisce un valore aggiunto; un valore aggiunto; e ciò per due ragioni. Innanzitutto, quel che si guadagna e si conquista viene ad avere una maggiore solidità perché quel risultato è meno esposto a ritorni indietro; in secondo luogo, vi è la possibilità per le donne di fare esercizio dell'autonomia, un grande principio che i maschi non sempre riescono a riconoscere e che è un valore per tutte le donne, quale che sia lo schieramento cui appartengono. anche piacere che diversi uomini abbiano accettato di sottoscrivere l'ordine del giorno, perché per dare attuazione agli impegni che il Governo si assume anche la loro cooperazione è importante. ricordare solo alcuni punti del dispositivo, che è molto articolato e ricco. Vorrei mettere al primo posto quello che qui compare all'ultimo semplicemente per un ordine logico. dell'impegno del Governo ad elaborare una proposta di codice di autoregolamentazione che fornisca linee guida al sistema radiotelevisivo perché si arrivi al massimo rispetto della rappresentazione della figura femminile. un altro impegno importante: quello di tenere adeguatamente in conto, in sede di stipula del contratto di servizio 2010-2012, i principi espressi nel parere della Commissione di vigilanza RAI.

iniziative legislative per dare attuazione alle direttive dell'Unione europea, oppure la valorizzazione di altri modelli di altri modelli di donne quelle che arrivano a conquistare posizioni nel mondo della cultura, delle professioni, dell'arte e della scienza. Allora, siamo davvero tutte convinte - per questo siamo riuscite a raggiungere questo risultato - che ci sia un grande problema nel nostro Paese nel rapporto tra donne e *media*. Le donne hanno risonanza nei *media* solo se sono vittime o veline: quindi non emerge adeguatamente quella figura di cui parlavo prima, che pure è così diffusa, anche se non come dovrebbe, nella società. C'è piuttosto invece il modello del successo facile, del diventare famosi ad ogni costo. Abbiamo richiamato molto opportunamente nelle premesse anche il monito del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, quando ha invitato a non fare un uso consumistico della donna e a non considerarla come oggetto.

anche sul piano simbolico. Quindi, ringrazio davvero tutte le colleghe, maggioranza e opposizione, e il Governo per aver tutte cooperato a raggiungere questo risultato.

così come è riportato il fatto che il Governo si è impegnato al momento della stipula del contratto di servizio a che questi principi appunto si traducano in quell'atto che mette d'accordo il Governo da una parte

unitario, condiviso dopo un proficuo confronto; è la chiara dimostrazione che con un po' di buona volontà, se si crede in un progetto, si può raggiungere un'intesa.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Ministro, la scorsa settimana ci siamo lasciati dicendoci che sarebbe stata un'occasione mancata non arrivare, su un tema del genere, ad una grande convergenza. Tutti i Gruppi si sono resi disponibili a questo tentativo di condivisione su un tema che - ripeto - è delicato e complesso per il nostro Paese, per la dignità delle donne e per il futuro delle generazioni. Abbiamo lavorato senza pregiudizi ad un ordine del giorno unitario, perché spaccarsi su quali sono le cause dello sfruttamento del corpo femminile nei *media*, avrebbe offeso in modo particolarmente grave le donne italiane. Vorrei ringraziare tutte le colleghe per il lavoro svolto e il ministro Carfagna per l'attenzione mostrata nell'accogliere le proposte di tutti i Gruppi. II testo a cui giungiamo oggi è frutto di una mediazione in cui, inevitabilmente, ognuno rinuncia a qualcosa del proprio progetto iniziale, in cui le premesse restano in alcuni punti generali e gli impegni, in alcuni tratti, meno cogenti. Badate, non è una critica, perché tutti sappiamo che nel momento in cui si cerca una soluzione condivisa, non potrebbe essere diversamente. Ritengo, anzi, che il testo che votiamo è innanzitutto la dimostrazione che quando le donne collaborano ad un progetto comune, e soprattutto credono in tale progetto, sono in grado di pervenire sempre ad un'intesa. Non mi soffermerò ad approfondire il problema del ruolo delle donne nei *media* e nella pubblicità, perché lo abbiamo esaminato abbondantemente la scorsa settimana e ognuno di noi si è espresso al riguardo. Ritengo infatti che sia chiaro a tutti che un intervento del Parlamento e del Governo sia ormai necessario e non più procrastinabile. Questo di oggi è un primo passo in tal senso. Affrontare il tema della distorsione degli stereotipi femminili nel mondo della comunicazione, in una società come la nostra, è un punto fondamentale. Ci è stato chiesto dall'Unione europea e dal Comitato CEDAW in seno all'ONU. Soprattutto ce lo chiedono tutte le dorme e gli uomini, disgustati da immagini pubblicitarie che riducono le stesse donne ad oggetti; da programmi televisivi in cui la componente femminile non conduce, non canta, non balla, ma è solo arredamento della scena. Non sono queste le cose che vogliamo vedere né ora né mai. Nella vita di tutti i giorni, le donne vere sono quelle che lavorano e studiano, che cercano di costruirsi una carriera, spesso tra mille difficoltà. È a loro che dobbiamo il massimo rispetto ed è per loro che dovremmo cercare, ancora una volta tutti insieme, di elaborare proposte concrete. Mi riferisco a misure che permettano di usufruire di forme lavorative flessibili, sia per quanto riguarda l'orario di lavoro che l'organizzazione del lavoro stesso, di sostegno alla maternità, di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita. Sono tutte cose già da tempo previste per legge, ma che ancora stentano a decollare: penso solo alla banca del tempo e al telelavoro. Mi piacerebbe che su questi temi che ho appena ricordato si potesse lavorare nuovamente insieme. Spero che lei, signora Ministro, voglia accogliere il mio invito. Mi avvio a concludere ribadendo che oggi, in quest'Aula, abbiamo ottenuto risultati positivi in termini di crescita sociale e culturale del nostro Paese, prima approvando un provvedimento che garantisce l'equilibrio dei generi negli organi di amministrazione delle società quotate e, ora, chiedendo che si ponga fine alle discriminazioni che sistematicamente i *media* operano nei confronti delle donne. In questi giorni in cui ricorrono i 150 anni dell'Unità d'Italia mi piace ricordare ciò che diceva Anna Maria Mozzoni, pioniera del femminismo italiano, negli anni in cui «fatta l'Italia bisognava fare gli italiani» e le italiane:

di incorrere in questo ritardo. Certamente ritiro la mia mozione, sulla quale comunque c'era stato il parere favorevole del Governo; ben volentieri ho sottoscritto questo testo che è stato presentato dalle colleghe senatrici di tutti i Gruppi, perché in realtà l'obiettivo di tutti è comune. È evidente che le premesse possono essere diverse, possono esserci delle diverse

Donne che però non siano soltanto brave giornaliste o brave inviate di guerra, ma che possano operare anche nei luoghi decisionali, proprio per indirizzare le

attraverso le parole di altri: altri parlano delle donne, non sono loro a parlare direttamente. È un'immagine femminile che spesso appare ed è in risalto per fatti tragici, più che per le capacità e la professionalità, come abbiamo detto anche nel corso del dibattito precedente.

crescita della pubblica opinione e promuova la ricerca di una nuova sintesi, che garantisca l'effettiva parità di genere come contributo per la crescita del Paese in termini di inclusione, coesione sociale e progresso culturale.

di una donna, di un essere umano, passa sempre attraverso il rispetto, in primo luogo, della sua dignità e della sua complessità.

stiamo promuovendo e su cui stiamo dibattendo in questi giorni ed è importante che le iniziative parlamentari sul tema delle donne siano siano accompagnate dal più ampio consenso possibile. Non dispero: ci sono stati grandi cambiamenti negli ultimi anni

il lavoro svolto al riguardo dal Governo mi pare vada nella la direzione giusta. Ho la sensazione che la pazienza delle donne, come racconta anche il bel testo di una canzone, cominci a produrre quell'elemento culturale

un principio che non può che far bene alla società e, quindi, a ciascuno di noi.

e compongono un *puzzle* fortemente negativo. Voglio qui brevemente ricordarne alcuni. In primo luogo, la globalizzazione, unita alla crisi economico-finanziaria, sta erodendo l'identità, le radici storiche e culturali, le tradizioni, il senso di appartenenza alla comunità, al territorio in cui si vive: valori che nei decenni scorsi hanno consentito la costruzione di un Paese di un Paese civile, in grado di essere motore di benessere e di crescita di una società sana; valori che guidano alla consapevolezza che ogni cittadino deve restituire alla comunità azioni che favoriscano il bene comune; valori che afferiscono al rispetto della dignità della persona indipendentemente dalle differenze di genere. Il tassello numero due è rappresentato invece dalla comunicazione multimediale, in grado di offrire una molteplicità di informazioni e saperi disponibili a tutti. È uno strumento positivo di liberazione culturale, e insieme uno strumento di controllo sociale, veloce, semplice ed esteso. La caduta sociale dei valori che afferiscono al rispetto della dignità della persona, in particolare delle donne, che vengono presentate attraverso stereotipi sminuenti e mercificanti, è amplificata inevitabilmente dalla comunicazione multimediale che replica così il relativismo, presentandolo come modello sociale da seguire. Terzo tassello. Se da un lato è chiara la responsabilità di chi gestisce i contenuti della comunicazione multimediale, dall'altro la Lega Nord non esita a prendere atto e a ribadire che buona parte dei contenuti negativi che afferiscono alla figura femminile sono accettati e, a volte, plauditi da un vasto pubblico, impreparato ad esercitare la capacità di riflessione critica nei confronti dei contenuti stessi, subendoli più o meno consapevolmente ed abbeverandosene. Quarto ed ultimo tassello. Non dimentichiamo che le donne stesse, per svariati motivi, accettano di interpretare ruoli stereotipati, di mercificazione La Lega Nord non vuole essere bacchettona, giudicando le scelte personali, ma non può esimersi dal porre in evidenza, senza ipocrisie, che questa è la realtà. Insieme, questa mattina, abbiamo saputo individuare azioni e proporre progetti al Governo, al fine di superare le connotazioni negative che riguardano i messaggi comunicativi, espliciti ed impliciti, sulle donne. In modo particolare, la Lega Nord ritiene indispensabile promuovere ogni iniziativa utile a valorizzare e potenziare gli strumenti di educazione dei giovani, ad un utilizzo critico, consapevole e responsabile dei mezzi Voglio qui ricordare che i nostri giovani sanno usare i mezzi di comunicazione ma non ne sanno comprendere i codici di linguaggio, mentre le loro famiglie, i loro genitori molto spesso non sanno nemmeno usare i mezzi di comunicazione. comunicazione. Altrettanto importante è la promozione del doppio ruolo della donna, quello all'interno della famiglia e quello nell'ambito del mondo politico, economico, culturale e scientifico. Famiglia, come sancita dall'articolo 29 della Costituzione e quale elemento fondante e primario per la crescita della società; opportunità, seguendo il principio del merito, della valorizzazione delle competenze, delle conoscenze e del riconoscimento della forza costruttrice delle donne, per quanto riguarda tutti gli ambiti professionali e politici. Forza che va sostenuta dalle istituzioni *in primis*, ma della quale devono esserne consapevoli le donne stesse. La Lega Nord ritiene che le donne debbano sentirsi orgogliose di essere donne e debbano essere valorizzate anche quando liberamente decidono di optare solo per la cura della famiglia, perché anche questo è importante per la crescita della società. Ringraziando le colleghe senatrici ed il ministro Carfagna per aver saputo esprimere un ordine del giorno snello, ma non per questo meno importante, esprimiamo, come Gruppo della Lega Nord, un voto favorevole al testo di quest'ordine del giorno e, proprio nella

PROCACCI *(PD)*. Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico ha voluto che fosse un uomo a tenere la dichiarazione di voto, perché la questione che stiamo affrontando non riguarda solo un genere, ma entrambi, e lo dimostrerò. È infatti una questione che tocca anche il nostro modo di essere uomini, di vivere e concepire il rapporto con l'altro genere. Occorre partire dalla constatazione che l'educazione e la formazione dei cittadini sono state in larga parte sottratte alla famiglia e alla scuola dai *media* e in particolare dalla televisione, che entra indisturbata nelle case di tutti gli italiani. Dunque, lo Stato non può limitarsi a prenderne atto, ma deve sentire su di sé il peso e la responsabilità di vigilare, e non solo sulla RAI, a che questo dato non si trasformi in un peggioramento e in una distorsione della formazione dei cittadini. Il 60 per cento delle immagini televisive è costituita da donne; quindi, non siamo dinanzi ad un problema di quantità, bensì di qualità. Infatti, si dà l'impressione che solo una certa bellezza sia strumento di successo, senza considerare altre qualità.

con prevalenza di primi piani su particolari anatomici e con telecamere, già prima della trasmissione, posizionate in modo da carpire immagini del genere, in una logica fondata sulla netta prevalenza dell'apparire rispetto all'essere. Questa continua rappresentazione della donna come oggetto sessuale crea modelli ed induce tante ragazze a ricercare il successo nei diversi campi, aggiustando ossessivamente il proprio corpo e smarrendo il diritto-dovere alla autenticità, alla verità, che si vive nella vita di ogni giorno, alla capacità di riconoscere i propri veri bisogni; quella rappresentazione produce anche tanta sofferenza a chi non può competere con quello strumento. Anche quando le donne vengono chiamate in TV per motivi professionali e per proprie competenze, non si rinuncia ad una logica che induce a guardarle con occhi - lo dico da uomo - maschili. Basti pensare a trasmissioni come «L'isola dei famosi» - dobbiamo avere il coraggio di affermarlo in questa sede - per comprendere immediatamente quanto poc'anzi affermato. Signora Ministro, quando ho personalmente chiesto al presidente della RAI come sia possibile mandare in onda certe trasmissioni, mi sono sentito mi sono sentito dire: «Anch'io un po' mi vergogno, ma sa quanto rendono in pubblicità?» La RAI purtroppo perde ogni anno il 25 per cento di canone non pagato dagli italiani. Inseguiamo dunque la logica dello *share* e delle televisioni commerciali, che la RAI talvolta finisce per imitare sottoponendosi alla dittatura della pubblicità e dell'*audience*... al punto che su Raidue qualche tempo fa, in una trasmissione, è apparso un tabellone elettronico su cui sarebbero comparsi i numeri di una ricerca statistica

calendario?». Signora Ministro, non si tratta di demonizzare la bellezza, come qualcuno in modo spregiativo sostiene, né di una visione moralistica di retroguardia, bensì di prendere atto del danno culturale, umano ed educativo che si produce alle donne e a tutta la società. Se infatti consideriamo i risultati del comitato TV e minori del 2004, ci rendiamo conto più facilmente che questo modo di ritrarre la donna in TV, ma anche sulla carta stampata (e non parliamo poi di Internet), produce gravi danni alle bambine che sono indotte a seguire modelli sbagliati,

Da questo *humus* nascono episodi di violenza sessuale, che non è solo quella che finisce nelle cronache, ma è anche quella che si consuma nel silenzio delle mura domestiche. Care colleghe e colleghi, votare questa mozione non significa soltanto affrontare una questione di pari opportunità e di rispetto per la dignità delle donne - pur obiettivi di per sé assai rilevanti - ma significa soprattutto comprendere che è in gioco qualcosa di più grande, che riguarda l'intera società italiana e che è l'educazione al giusto rapporto tra i generi, l'educazione all'amore come fondamento di un ordine sociale migliore, capace di elevare il livello civile del nostro popolo. Occorre avere il coraggio di affermare che l'amore (parola difficile da pronunziare in Parlamento) come dimensione fondante della persona umana è un fatto privato nel suo vissuto individuale, ma nella dimensione educativa è un fatto pubblico, di cui lo Stato e la politica devono farsi carico anche se sappiamo che su questo aspetto lo Stato e le sue agenzie formative (a cominciare dalla scuola) sono latitanti, forse perché erroneamente credono che non sia compito loro. Ma chi crede nel valore della famiglia e nella sua centralità, chi auspica una società più giusta e meno violenta, deve essere consapevole che questi obiettivi si perseguono soprattutto educando i cittadini ad una sana affettività, ad una capacità di amare che sappia andare oltre la pura corporeità (che è di per sé un valore, ma non sufficiente), che sappia coniugare la bellezza con la tenerezza, che sappia cogliere la bellezza non solo nella fisicità, ma anche nel fascino straordinario della identità altra da sé. Come ci si può nascondere che la mancanza di questa capacità di amare e l'inseguire questi modelli distorti che i *media* ci propinano è una delle ragioni più frequenti che portano alla dissoluzione delle famiglie e alla conseguente diffusione della violenza? Ma chi educa all'amore nel nostro Paese? La famiglia? Poco o mai! La scuola men che meno! Dunque il Parlamento affronti questa questione: è una questione nuova, signora Ministro. Impostare la questione delle pari opportunità sulla radice più profonda di un aiuto e di una tutela di un genere soltanto è un'idea secondo me fondamentale anche per le sue politiche di Governo. Il Parlamento, dicevo, affronti questa questione perché è compito dello Stato, secondo me il quale, non solo non educa, ma al contrario, consente, non vigilando, una profonda distorsione della dimensione formativa. Vorrei che tutti i parlamentari (l'ha già richiamato qualche collega) potessero vedere quel documentario

Al modello di donna nelle TV di oggi, che ha vergogna per ciò che il tempo ha naturalmente prodotto sul volto, quel documentario oppone Anna Magnani, che sul *set* di un film dice ad un affannato truccatore: «Non cancellarmi nemmeno una ruga, ci ho messo tanto tempo a farle!». Mascherare il volto, omologandolo ad uno stereotipo, significa rinunciare al fascino della sua vulnerabilità, alla sua identità, alla sua espressività e soprattutto alla sua irripetibile unicità! Da tutte queste considerazioni nasce l'invito al Governo ad impegnarsi perché siano rispettate tutte le risoluzioni, nazionali ed europee, che impegnano i *media* ad adottare e rispettare un codice di autoregolamentazione che tuteli la dignità della donna.

Chiudo, perché il tempo è tiranno. Voglio soltanto dire che è importante e significativo che su questo tema oggi si voti tutti la stessa mozione. È un segno di unità su un grande tema che riguarda la convivenza civile del nostro Paese. Tutto questo rafforza il mandato che il Parlamento dà al Governo e agli organi preposti alla gestione della comunicazione. Questa unità di intenti è stata raggiunta grazie all'impegno di tutti i Gruppi parlamentari, ma - devo dirlo - soprattutto delle senatrici (altro che divisioni per colori: quando si uniscono sono una potenza della natura!), che non si sono arrese a quella che sembrava una ineluttabile contrapposizione. Ma consentitemi di dire questo: il felice esito di questa mozione è stato possibile anche perché - vorrei fosse dato atto di questo - il Partito Democratico non ha usato parole sul cui sfondo potessero materializzarsi fantasmi di cronaca attuale. non ne abbiamo parlato, né abbiamo parlato di comportamenti di uomini pubblici che alimentano questa subcultura, e non intendiamo farlo! Sarebbe persino facile! Ma sarebbe anche l'ultima beffa per le donne, perché renderebbe falsa, inautentica e strumentale una battaglia che invece vuole essere per l'autenticità, la verità e per la dignità della persona umana. *(Applausi

Networks* ha un ruolo crescente nella vita delle persone con nuove opportunità e nuovi rischi, richiedendo alle tradizionali agenzie educative una maggiore e diversa responsabilità e presenza per contrastare

la favorevole circostanza che oggi non sia 1'8 marzo e si parli di donne e di riconoscimento di ruoli, di protezione di dignità e di pubblica immagine, di affermazione paritaria di preziose diversità, di pari opportunità in senso proprio, propositivo e concreto, sgombra definitivamente il campo all'ingenua associazione del tema a stantie rivendicazioni sessiste e lo pone, viceversa, nella giusta prospettiva. Pretendere oggi che la rappresentazione dell'universo femminile comunemente data dai mezzi di comunicazione, e quindi percepita, corrisponda al vero è, da una parte, la naturale ed equilibrata continuazione di quelle prime infuocate battaglie; dall'altra, l'espressione più moderata, saggia e onesta del recupero del mezzo di comunicazione come agenzia educativa e di formazione delle nuove generazioni. Mentre in Italia le donne lavorano con pari diritti dell'uomo, si affermano nello studio, nelle professioni, nell'imprenditoria, nell'arte, nella cultura, nel sociale, nel sindacato; dopo decenni di battaglie per ottenere visibilità e ruolo nelle istituzioni; dopo aver penetrato realtà lavorative impenetrabili come, ad esempio, quella militare o della magistratura; dopo aver fatto emergere realtà familiari fatte di violenze e prevaricazione e aver cercato e trovato soluzioni normative e di contrasto che fanno scuola; dopo aver rivendicato l'importanza della bigenitorialità all'interno della famiglia; dopo esserci poste in prima linea nel mondo a fianco di tutte quelle donne che questi diritti non hanno e sono ben lontane dall'ottenerli; ebbene, dopo tutto questo, il rischio è che, nei pochi minuti dei telegiornali o nelle lunghe ore di *fiction*, *reality* e *talk show*, nei «6 per 3» pubblicitari o nelle copertine dei *magazine*, la donna sia rappresentata, e quindi, ahimè, idealizzata, come rispondente ad uno stereotipo che non corrisponde allo spaccato della società italiana: che non è poi così violenta, inoperosa e faceta; che viceversa è fatta di normalità, di quotidianità, di bellezza e giovinezza che sfioriscono, di ricchezza ma anche di sacrificio; di donne che conciliano la naturale vocazione alla maternità con il proprio lavoro. Dico idealizzata perché il passaggio dalla falsa rappresentazione di un modello alla credibile strutturazione sociale dello stesso è quasi automatico. È il fenomeno crescente e tristemente noto di adolescenti che desiderano carriere rapide nel mondo dello spettacolo, legate più all'effimero e all'apparire che a una professionalità e a una preparazione culturale. Sarebbe poco se il problema consistesse solo nella sovraesposizione mediatica e volgare del corpo femminile. È molto peggio. È molto di più. C'è il problema di fondo, e assai più grave, della violenza verbale, di immagini e stereotipi con cui lavora quotidianamente l'informazione. E dire che va dato atto alla TV e non solo pubblica, come riconosciuto anche dall'Unione europea di aver dall'Unione europea di aver messo in campo, negli ultimi anni, un tentativo di porre all'attenzione del pubblico donne protagoniste di storie di vita ordinaria o straordinaria che fossero modelli positivi e avessero come filo conduttore un profilo valoriale forte e inequivocabile. Tra le più recenti ricordo Maria Montessori, ad esempio, con il suo coraggio e la sua pedagogia che precorre i tempi; Edda Ciano che rivendica il diritto di innamorarsi di un comunista; le sorelle Fontana che, partite dalla provincia, realizzano con caparbietà e sacrificio i propri sogni creando un impero finanziario; «Butta la luna», che affronta il problema

Il problema c'è paradossalmente - come ha dimostrato l'indagine commissionata dal CENSIS - non quando scatta la narrazione e il racconto, ma quando le donne che abitano la TV (reclutate secondo criteri di *audience*) rappresentano se stesse e vengono individuate come soggetti che fanno opinione. Il problema del deterioramento dell'immagine femminile si aggrava ancora quando, nei circa 30 minuti di telegiornale, reiterato nell'arco della giornata in fascia non protetta e su tutte le reti, le donne sono: uxoricide o infanticide, vittime di stupri e violenze, *pusher* della droga, giovani ereditiere di anziani magnati; e altro ancora. Se conta la popolarità e non come la si è raggiunta si spiega anche perché Erika, Amanda Knox e perfino Sabrina Misseri, accomunate nel probabile o accertato ruolo di assassine, ricevono sostegno e proposte di matrimonio dai fan. Ecco, chiediamo che venga fatto un po' di ordine affinché bambine e adolescenti che crescono non si buttino nel Bengodi che non c'è; affinché non desiderino, per fermarci al problema estetico, la magrezza eccessiva come modello o prominenze conquistate a suon di bisturi; affinché non puntino al successo nella vita (che è un fatto positivo) senza contemporaneamente accettare la strada del sacrificio, dello studio e della selezione: in una parola della meritocrazia per conseguirlo. Forse, dico forse perché non sono certa che sia così prevalendo sempre la logica del mercato e dell'*audience,* se ci fossero più donne nei gangli del potere mediatico ne uscirebbe un quadro meno sconfortante. Ma è più probabile, invece, che dovranno proprio essere gli uomini a mettere fine a questa virtualità del mondo dell' immagine della donna che tanto li fa sognare ed esaltare. La femminilità della donna si nutre, in ogni momento della vita e della storia, della complementarità del ruolo che l'uomo intende giocare: uomini, questi di cui parliamo, che sono anche padri e fratelli e dovranno alla fine percepire il problema. Cioè: se continuerà ad esserci domanda di oche in TV e di nudo sui giornali, sarà perché gli uomini preferiscono relazionarsi a queste categorie. Senza tirare in ballo enunciazioni filosofiche parmenidee o il concetto di complementarità uomo/donna, che assume volti diversi nella civiltà contadina o industriale, al Nord o al Sud, in ambienti cattolici o non, mi basta citare la simpatica frase di Bertold Brecht: che ne è dei buchi quando è finito Nei banchi del PdL siedono donne che nella loro vita per motivi anagrafici, scelta culturale o educazione familiare non sono scese in piazza a fianco di quelle femministe che rivendicavano prima di tutto la libertà sessuale e di esibizione del corpo e la liberazione da schemi asimmetrici che esprimevano, a parità di comportamenti, giudizi di valore e morali diversi. È stato, il nostro, un modello di rivendicazione poco eclatante, ma senza sosta: condotto in famiglia, a scuola, nelle università e nei luoghi di lavoro per farci valere, per avere innanzi tutto l'indipendenza economica, per prenderci ciò che non volevano darci. Un femminismo parlato e non urlato, strisciante (se così lo si può chiamare), che faceva moderata eco a ciò che succedeva in strada, e che leggevamo nei libri e sui giornali. Siamo pronte oggi a riconoscere quanto importante sia legittimare a vicenda, in un unico modello, gli obbiettivi e i risultati di quante allora scesero in piazza e di quante invece custodirono modelli più tradizionali, accomunate tutte, oggi, in un'unica equilibrata visione: quella di recuperare quel 50 per cento di «talento vero» di cui l'Italia ha assoluto bisogno. Ogni rivoluzione si traduce in una sintesi che segue il cambiamento: in fondo, a pensarci bene, il termine rivoluzione è mutuato dall'astronomia e vuol dire, riferito agli astri, faccio un giro e ritorno al punto di partenza. È un mutamento che comporta la rottura di un modello e il sorgere di uno nuovo; comporta, cioè, il ritrovare un nuovo equilibrio: per questo, colleghe, non possiamo permetterci che le infinite rivoluzioni femministe e femminili abbattano tabù e valori lasciando il vuoto davanti. Sarebbe folle non aver chiaro il nuovo quadro valoriale e sociale o, peggio ancora, non averlo affatto. Insomma: non abbiamo invocato libertà ed eguaglianza e detto che 1'essere madri non doveva impedirci di avere anche un'altro ruolo nella società per veder minimizzato alla fine, sia l'uno che l'altro. Come non ricordare allora quelle donne che 150 anni fa contribuirono in maniera decisiva a fare 1'Italia? La contessa Gambarana Frecavalli, che faceva la staffetta portava tra i capelli i messaggi che i congiurati lombardi si scambiavano con quelli del Regno di Sardegna; Bianca Milesi, allieva di Canova, pittrice amica di Hayez, che inventò la cosiddetta carta stratagliata, un foglio bianco con tagli orizzontali che permettevano di leggere messaggi segreti in testi apparentemente normali; la padovana Tonina Masanello, la quale, travestita da uomo, raggiunse i Mille in Sicilia per combattere con loro; Colomba Antonietta Porzi, la quale, tagliati i capelli e indossata la tenuta da bersagliere, seguì il marito in battaglia e morì a Roma: a lei è dedicato un busto al Gianicolo; Giuditta Tavagni Arquati, che aveva messo a disposizione dei patrioti la sua casa a Trastevere e, partecipando a una riunione, venne uccisa incinta del quarto figlio;

a Napoli insieme a Garibaldi; Cristina Trivulzio di Belgiojoso, intellettuale e femminista che contribuì ad organizzare le truppe a Napoli per le Cinque giornate di Milano. Non ho citato le più famose famose né quelle anonime, che però vanno ricordate e che hanno dato, direttamente o indirettamente, il proprio silenzioso contributo. Ecco, con il nostro convinto sì alla mozione sì alla mozione ci aspettiamo che vengano raccontate queste storie e l'anima che c'è dietro e che venga garantita nei *mass media* l'immagine più genuina delle italiane e quel patrimonio di valori, di conquiste e di diritti che orgogliosamente ci appartiene. E sommessamente auspichiamo anche che a rappresentare in TV le nostre idee e il nostro lavoro, accanto alle bellissime e bravissime deputate d'acciaio, appaia, talvolta, anche qualche collega meno bella e più fragile, magari con qualche ruga di troppo e qualche dubbio in più. Insomma, per come intendo io la femminilità, più donna. Che cos'è poi la femminilità? Rispondo, e concludo, citando la poetessa, artista e intellettuale futurista Valentine de Saint Point che, replicando al misogino Marinetti dice nel manifesto della Donna Futurista il 25 marzo 1912, cioè 99 anni fa: «È assurdo dividere l'umanità in donne e uomini; essa è composta soltanto di femminilità e di mascolinità (...). Ogni donna deve possedere non soltanto delle virtù femminili, ma delle qualità virili; altrimenti è una femmina.

devo intervenire su una questione tecnico-giuridica piuttosto delicata, con evidenti risvolti politici, che è stata richiamata in quest'Aula, anche oggi pomeriggio, *incidenter tantum*,

sia in ambito giornalistico, è stato fatto riferimento alla posizione assunta dal Senato a questo proposito in una precedente vicenda relativa all'allora ministro Mastella. Preciso subito che si tratta di una fattispecie molto diversa, di un caso giuridico molto diverso rispetto a quello che dovrebbe condurre domani, alla Camera dei deputati, a un conflitto di attribuzione tra magistratura e Parlamento. Siccome anche in quest'Aula il senatore Mazzatorta ha fatto riferimento alla decisione del Senato, che avrebbe attribuito al Parlamento la competenza sulla qualificazione giuridica, e siccome viene riportata questa posizione come unanime, sia in ambito parlamentare che all'esterno, desidero ricordare quella che invece era ed è la nostra posizione.

che su questo punto e sulla vicenda del conflitto di attribuzione, per i risvolti politici che avrà, sia competente a decidere, non il Parlamento, ma la magistratura. Quindi, la qualificazione della natura ministeriale

compete, a nostro modo di vedere, alla magistratura e non al Parlamento. Tanto ritenevamo allora e tanto ribadiamo questa sera.

Signor Presidente, desidero riferire alla Presidenza e all'Aula di un fatto che tocca nella tragedia del Giappone la nostra precisa responsabilità parlamentare e di Governo.

Vi è stata troppa incertezza nella decisione del rientro, come se non fosse prioritaria la scelta per la sicurezza e la salute di fronte ad altri interessi pur legittimi culturali, economici e politici. Vi sono state pressioni psicologiche all'inizio perché non rientrassero. Non mi risulta fino a questo momento che il Governo abbia riconosciuto l'emergenza mettendo quindi prontamente a disposizione i mezzi necessari perché potessero lasciare immediatamente il Giappone. Ogni ora che passa la situazione peggiora: le scosse, il panico e il rischio nucleare sono gli ingredienti di una dimensione esistenziale di vita di queste ore che è gravissima. Chiedo alla Presidenza che solleciti il Governo perché immediatamente provveda e perché venga anche in quest'Aula a dar conto di questa vicenda particolare nella tragedia del Giappone che ha colpito l'umanità l'umanità intera e anche noi. Su questo punto specifico è nostra responsabilità, del Governo e del Parlamento, fare in modo che siano messe in sicurezza le persone del Maggio musicale fiorentino sono là e hanno dato prova, nonostante le difficoltà psicologiche, di grandissima umanità e professionalità realizzando fino a pochi giorni fa gli spettacoli che sono stati commoventi per tutto il pubblico giapponese.

Concordo anche nel merito con le considerazioni che ha fatto. Credo anch'io che ci sia stata una decisione tardiva e sbagliata sul rientro perché in queste situazioni il il primo punto è quello di garantire la sicurezza delle persone: non c'è dubbio. Questo è un elemento che esiste. Oggi c'è una necessità su cui la Presidenza interverrà per sollecitare il Governo perché siano messi

facoltà. VIMERCATI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per stigmatizzare e chiedere alla Presidenza del Senato l'intervento presso il Governo per quanto è avvenuto questa mattina nell'aula del Consiglio regionale della Lombardia.

perché l'inno di Mameli, così come la bandiera, rappresenta tutti noi, tutti gli italiani, tutti i lombardi. Credo che questo sia un insulto anche ai tanti lombardi che - non dimentichiamolo - sono eredi di quei Mille che hanno fatto l'Italia. Tra quei Mille c'erano 180 bergamaschi, decine di pavesi e di varesini, di milanesi, di bresciani e così via. Credo che questo sia un insulto inaccettabile. Proprio questa ragione credo sia importante stigmatizzare quanto è avvenuto. Credo che la pezza che ha voluto mettere il presidente Formigoni sia, se possibile, peggio. Quando il presidente Formigoni a commento ha detto che 70 secondi dell'inno di Mameli non fanno male a nessuno, ha dato l'idea che l'esecuzione dell'inno è un mero fatto burocratico, di *routine*, non un momento alto per un Consiglio regionale come quello della Lombardia. Per queste ragioni, chiediamo come Partito Democratico alla Presidenza del Senato di stigmatizzare quanto è avvenuto e di chiedere al Governo

sulla Costituzione, sulla bandiera e sull'inno. E sul fatto che questo Paese può fare, come dice il Presidente della Repubblica, tutte le riforme (federalismo ed altro) a partire da questi aspetti.

del personale volontario dei Vigili del fuoco, senza nulla togliere naturalmente ai Vigili del fuoco, che il Partito Democratico ha sempre difeso, perché hanno una carenza di organico veramente importante. Si tratta di porre l'attenzione, per non disperdere le competenze, su persone che hanno un bagaglio tecnico e professionale acquisito con un percorso formativo. Chiedo perciò al Ministro e a lei, signor Presidente, di farsi parte attiva per salvaguardare queste figure che vanno a completare un processo di immissione in ruolo di coloro che oggi sono in una graduatoria di stabilizzazione. Domani queste persone, volontari dei Vigili del fuoco, pacificamente manifesteranno per l'ennesima volta davanti a Montecitorio. Ecco, vorrei che venissero prese in considerazione.

hanno bloccato l'autostrada Palermo-Catania, visto che, dopo le bugie di Scajola, le pacche sulle spalle del ministro Romani non sono servite a risolvere il problema gravissimo dello stabilimento. è il rischio di perdere il lavoro, non solo per quegli operai ma per tutto l'indotto attorno allo stabilimento di Termini Imerese: famiglie, che aspettano ancora il piano industriale, così come è stato promesso dal Governo Berlusconi, da Scajola prima e dal ministro Romani adesso. Ecco perché chiediamo che il ministro Romani venga a relazionare

che altro non fa che togliere lavoratori per metterne altri. che il loro patrimonio professionale venga tenuto in considerazione e che non venga sottovalutato il problema sociale che deriverebbe dal loro proclamato ed imminente licenziamento. Che cosa vuole fare Trenitalia? licenziare 500 persone nel comparto dei treni notturni, in concomitanza con le centinaia di assunzioni che la stessa Trenitalia ha stabilito e sta già effettuando per fare fronte all'incremento occupazionale previsto per i treni con percorrenza diurna:

visto che stiamo parlando di perdite di posti di lavoro, di garantire una tutela di queste persone, che hanno mutui da pagare, famiglie da mantenere, che vogliono portare ancora a scuola i loro bambini e poter mangiare. Questa è una sollecitazione che farò al Ministero, ma che rivolgo anche alla Presidenza, perché parliamo